ad un membro della nostra Giunta delle elezioni, riguardanti un presunto recupero di 8.007 voti da parte dell'Unione nel riconteggio delle schede. Al riguardo, vorrei precisare che il Regolamento prescrive la segretezza e la riservatezza sui dati della revisione

Presidente, non so che cosa i giornalisti abbiano capito di quello che un nostro collega senatore ha detto loro sul lavoro dei sette comitati che stanno rivedendo le schede bianche e nulle. Un fatto è certo: basta che il collega Malan, come tutti i colleghi

i conteggi effettuati fino alla settimana scorsa e a verificare se c'è un segno più o un segno meno. Questo per dovere di correttezza. *(Commenti

di segnalare che nei lavori dei seggi vige una regola di riservatezza, se non di segretezza. La Giunta per le elezioni, nella stragrande maggioranza dei suoi componenti, ha preso atto che non risultavano anomalie rilevanti dall'esame delle schede bianche, nulle e contestate fino ad oggi effettuato e ha deciso di sospendere per un attimo, alla percentuale del 25 per delle schede bianche, nulle e contestate e di avviare (secondo una delibera che già precedentemente era stata assunta) l'esame delle schede valide. Abbiamo già provveduto, attraverso i nostri Uffici, a richiedere ai tribunali competenti l'invio dei plichi e quindi quanto prima cominceremo l'esame delle schede valide. Per quanto riguarda i conteggi e i numeri che sono stati dati, penso che il presidente Nania in una delle prossime riunioni della Giunta farà il punto della situazione, certamente quando avremo raggiunto la soglia del 25 per cento, e quindi si avrà contezza dei numeri esatti evitando di dare i numeri al Lotto.

è, innanzitutto, da constatare la violazione, se vi è stata, di un dovere istituzionale di riservatezza da parte di un nostro collega. Mi auguro ancora che non si tratti di questo e spero che dal collega Casson venga rapidamente, magari in quest'Aula, una smentita di quanto abbiamo letto sui giornali e a lui attribuito.

La seconda questione, ancora più grave, è che, nel momento in cui si viola questo dovere di segretezza, lo si fa diffondendo una notizia falsa che, come è noto, diventa poi la notizia e a nulla valgono le smentite che noi ieri abbiamo indirizzato agli organi di stampa, senza però violare la riservatezza sui numeri. abbiamo detto soltanto che ci auguriamo che quello che abbiamo letto non sia da attribuire al collega Casson e che comunque le cose non stanno così, oltre non siamo andati. qualche minuto fa il collega Lusi ha voluto ribadire il concetto, sbagliato, che i giornali hanno attribuito al collega Casson, cercando di strumentalizzare ancora una volta questa vicenda. Anche il collega Boccia è incorso in qualche modo in una imprecisione. La Giunta non ha deciso di sospendere perché non ha rilevato anomalie:

invece che la verifica delle anomalie doveva attuarsi in questa fase sulle schede valide e che, stante i tempi tecnici per richiedere le schede valide alle corti d'appello, che non sono indifferenti, doveva predisporre i campioni per poter procedere a questa richiesta, profittando anche di questa fase di sospensione data l'inagibilità per la prossima settimana della sala Koch. Lei sa, Presidente, che la questione è delicatissima e attiene alla legittimazione stessa di tutti noi in Aula. Noi che dall'opposizione abbiamo per primi, dal giorno delle elezioni, chiesto il controllo, ci siamo attenuti a rigorosi criteri di silenzio nei confronti della pubblica opinione, anche quando giungemmo al risultato, per noi auspicabile e desiderato, di convincere l'intera Giunta per le elezioni, l'intero Senato a procedere a questa revisione ed a ciò seguì la decisione della Camera. La prego di intervenire, con la fermezza che le è propria ed abituale e con il rispetto delle regole che lei non ha fatto mai mancare, perché non si abbiano a ripetere atti simili e perché - questo mi sembra fondamentale

di rispettare le regole della formalizzazione prima di diffondere atti, prenderò contatto direttamente con il presidente Nania. Aggiungo, sul piano più generale, che il tema e le considerazioni fatte per primo dal senatore Malan toccano un problema più ampio, che in qualche modo deve essere governato nel rapporto tra decisioni formali e organi di stampa, che stanno creando, proprio in queste ore, ulteriori problemi che toccano la sensibilità del Paese.

presentata riguarda un argomento specifico delle politiche ambientali del nostro Paese, che però è essenziale per poter informare di sé

con occasioni anche di nuova occupazione. Il punto è: quali sono le politiche per affrontare la drammatica questione dei mutamenti climatici? I mutamenti climatici non sono più soltanto una minaccia per il futuro del pianeta, ma una realtà che interessa ormai anche le nostre latitudini, come dimostrano i fenomeni sempre più estremi che si succedono in Europa e nel Nord America, penso alle alluvioni, ai tifoni, anche ai lunghi periodi di siccità, come ad esempio quello che in questa stagione e che già sta suscitando un gravissimo allarme nel bacino del Po. Certo, resta il paradosso per cui a pagare il prezzo più alto di tali mutamenti sono quei popoli che non hanno alcuna responsabilità nell'aumento dell'effetto serra, a partire da ciò che succede nell'Africa sub-sahariana dove milioni di uomini e donne sono profughi ambientali costretti a spostarsi dall'avanzamento della desertificazione. Ed ormai sulla correlazione fra questi mutamenti climatici, l'aumento dell'effetto serra e le attività antropiche (la produzione di energia e i trasporti innanzi tutto) la comunità internazionale ha raggiunto un quasi unanime accordo, come dimostra anche la recente Conferenza dell'IPCC di Parigi. Allarmi che suscitano gravi preoccupazioni al punto da ritenere che siamo davanti ad un'emergenza ambientale mai vissuta da questo pianeta nel passato. D'altra parte, siamo convinti che la necessità di procedere a importanti cambiamenti nel modo di produrre e distribuire energia, nelle modalità di trasporto di persone e merci, rappresenta anche una straordinaria occasione di modernizzazione del sistema economico, specialmente in un Paese come l'Italia, che ha bisogno di dosi massicce di innovazione anche per consentire alle proprie imprese di competere nel mondo dell'economia globalizzata. Per questo una delle sfide più importanti e impegnative che la politica oggi deve affrontare è quella di uno sviluppo sostenibile: uno sviluppo in grado di far fronte alle esigenze di migliore qualità ed equità sociale delle presenti e future generazioni, senza compromettere l'ambiente, il clima, le risorse naturali del nostro pianeta, valorizzando anzi la qualità ambientale come fattore cruciale del benessere economico e sociale. Ridurre fortemente la dipendenza dal petrolio e, in generale dalle fonti fossili, puntare sull'efficienza energetica e sulle energie pulite, rinnovabili e su modelli di produzione di energia diffusi sul territorio: ecco l'esempio migliore, più attuale, di un'azione riformista che, al tempo stesso, è indispensabile per rispondere a una minaccia ambientale incombente (un irreversibile e catastrofico cambiamento del clima globale), ma anche per favorire uno sviluppo economico più duraturo, più diffuso e tecnologicamente più avanzato. Una straordinaria occasione per l'innovazione e la modernizzazione ecologica del sistema produttivo. Il nostro Paese però, è noto, è in grave ritardo nel raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas serra previsti dal Protocollo di Kyoto. Questo Governo, con la sua prima finanziaria, ha segnato una decisa inversione di tendenza: ed è stata ad esempio varata una sostanziosa modifica della legislazione sull'efficienza energetica negli edifici. Il risparmio energetico è infatti la più importante politica industriale che dobbiamo mettere in campo per raggiungere tali obiettivi. Ora è decisivo intervenire nella legge delega sull'energia che stiamo attualmente discutendo in 10a Commissione per per cambiare i meccanismi di incentivazione delle fonti rinnovabili, estendendo a tutte (eolico, geotermico, biomasse, mini-idro) il conto energia attualmente in vigore solo per il fotovoltaico, meccanismo di incentivazione che ha dimostrato di funzionare bene in tutto il mondo e in grado di garantire finalmente un grande slancio di questo settore che, oltre ad essere decisivo nella lotta contro i mutamenti climatici, può fornire nuove occasioni di sviluppo e di occupazione. Credo non sia un caso se, per esempio, in Germania in questo settore ci sono circa 200.000 occupati. Inoltre, è assolutamente necessario semplificare le procedure autorizzative anche per impedire che sorgano nefasti effetti NIMBY (*not in my back yard*), persino nella realizzazione di impianti da fonti rinnovabili. Dobbiamo coinvolgere in ogni caso le Regioni e gli enti locali nel raggiungimento degli obiettivi che ci siamo dati sia in termini di diffusione delle stesse e, più in generale, di riduzione delle emissioni di gas serra. Proprio in un'ottica di politica di riforme che modernizzi il Paese e metta al centro lo sviluppo sostenibile, un' utile occasione da cogliere è quella offerta dalle liberalizzazioni in corso. Il 1° luglio 2007 entrerà in vigore la completa apertura del mercato elettrico alla concorrenza che da quella data interesserà anche la clientela domestica. La liberalizzazione del mercato può rappresentare anche una grande occasione per premiare l'efficienza energetica degli operatori e il risparmio domestico da parte delle famiglie: la revisione delle tariffe dovrà però permettere ai cittadini di scegliere tra offerte diverse e quindi di scegliere di acquistare energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili. Proponiamo, pertanto, di intervenire con nuovi provvedimenti legislativi che incentivino il risparmio dei consumi elettrici domestici, applicando tariffe ridotte in bolletta agli utenti che realizzano una diminuzione dei consumi pari ad almeno il 10 per cento rispetto all'anno precedente; consentano la scelta, da parte dell'utente, di fornitura di energia elettrica prodotta con fonti rinnovabili; incentivino la possibilità di una fornitura di energia elettrica certificata proveniente da impianti alimentati con fonti rinnovabili anche attraverso incentivi fiscali che premi la nascita di questi nuovi impianti; intervengano intervengano in modo che tutti gli utenti possano scegliere tra piani tariffari e fasce orarie che incentivino soprattutto l'efficienza energetica. Ma per cambiare davvero strada sul fronte delle emissioni non possiamo trascurare il settore trasporti, che contribuisce, in maniera decisiva, all'aumento dell'effetto serra. È proprio in questo settore che servono i cambiamenti più radicali anche dal punto di vista culturale, nei nostri stili di vita, di questa nostra civiltà fondata sull'automobile, ma anche sulle scelte politiche relative alle infrastrutture a livello nazionale e regionale: investimenti su ferrovie e autostrade del mare, non nuove strade e autostrade. Sarebbe questa una scelta strategica responsabile. Infine, è evidente che, parlando di mutamenti climatici, non possiamo non considerare la forte riduzione dei fenomeni piovosi e delle precipitazioni nevose che quest'anno pone, con estrema severità, il problema della disponibilità di acqua per i diversi usi. In particolare, gli ultimi dati a disposizione circa l'entità delle risorse idriche del bacino padano rilevano che, a fronte di una portata del Po già inferiore a quella registrata l'anno scorso in pari periodo, il manto nevoso disponibile ricopre meno di un terzo del territorio coperto nel febbraio 2006 e con altezze altrettanto ridotte. Se entro aprile non interverranno significative precipitazioni, ad oggi improbabili, la situazione potrà risultare estremamente critica. Occorre quindi, per quanto concerne le produzioni agricole, dare subito l'avvio ad un'azione sui sistemi irrigui che possa condurre a forti risparmi e serve, per il futuro, una programmazione agricola che tenga conto della scarsità della risorsa acqua. È comunque necessario dichiarare sin d'ora lo stato d'emergenza per il bacino del fiume Po e per i bacini limitrofi e indire al più presto una conferenza nazionale sull'acqua nella quale affrontare il problema complessivo dello squilibrio tra fabbisogni e disponibilità idriche aggravato dai mutamenti climatici in atto.

e, da questo punto di vista, è assolutamente decisivo organizzare nei prossimi mesi e al più presto possibile una conferenza sull'energia e sui mutamenti climatici che affronti entrambi gli argomenti al fine di fornire una prospettiva futura a questo Paese in cui lo sviluppo sostenibile non sia più solo una chimera ma sia invece l'asse fondante delle nostre politiche industriali. **Sul rilascio dei due

Signor Presidente, onorevoli colleghi, mitigare e controllare gli effetti del cambiamento climatico in atto è una delle sfide più importanti che abbiamo davanti: i mutamenti del clima possono infatti minacciare la prosperità, la stabilità, lo sviluppo economico della nostra società. I rapporti elaborati dagli scienziati dell'ONU in questi mesi

ancorché non sia chiaro quale sia l'incidenza effettiva di tali attività né possano essere completamente ignorate le pur autorevoli voci di segno contrario. In ogni caso, il Protocollo di Kyoto ci ha fornito gli strumenti per raccogliere la sfida, anche se deve ritenersi che il Protocollo non sia più sufficiente per arrestare l'aumento dei gas serra in atmosfera. Non è sufficiente perché gli obiettivi posti sono frutto di una difficile mediazione, non è sufficiente perché ne sono fuori Paesi industrializzati come gli Stati Uniti e Paesi emergenti come Cina, India e Brasile che sono e saranno i Paesi a più alte emissioni di anidride carbonica. Secondo il rapporto 2006 dell'Agenzia internazionale dell'energia, la domanda globale di energia primaria aumenterà del 53 per cento entro il 2030: per cento di questo incremento arriverà appunto dai Paesi emergenti con in testa Cina ed India. Secondo la stessa Agenzia, nel 2010 la Cina diventerà il primo Paese per emissioni di CO2superando gli Stati Uniti e da sola sarà responsabile, pertanto, del 39 per cento dell'aumento delle emissioni globali da qui al 2050. Questo scenario insieme agli ultimi rapporti ci sollecitano quindi ad agire con maggiore risolutezza, ma dobbiamo essere tutti consapevoli che, se si vuole affrontare il problema climatico in maniera credibile e pragmatica, occorre costruire già oggi una prospettiva per il dopo Kyoto che coinvolga una platea di Paesi la più ampia possibile. Occorre quindi uno sforzo a livello mondiale per stringere, da una parte, un patto ambientale per il dopo Kyoto con gli Stati Uniti, la Cina, l'India, il Brasile e le altre economie emergenti, affinché si pongano obiettivi di riduzione dei gas serra, e per disseminare, dall'altra, tecnologie a basso contenuto di carbonio nei Paesi in via di sviluppo. Il G8 Ambiente, che si è aperto a Potsdam in Germania con la partecipazione di Cina, India, Brasile, Sud Africa e Messico, può costituire un primo appuntamento per accelerare il coinvolgimento di questi Paesi nella platea del dopo Kyoto. Senza questi Paesi, infatti, non sarà possibile un dopo Kyoto. L'Europa può decidere di andare avanti, ma deve essere consapevole che la sua battaglia solitaria avrà un impatto di fatto minimale sul fronte dei cambiamenti climatici e un impatto insostenibile, purtroppo, sulla competitività del suo sistema produttivo. Il Vertice europeo della scorsa settimana ha approvato un Piano di azione energetico per mitigare e controllare gli effetti dei cambiamenti climatici legati all'attività umana che ha, tra i suoi punti qualificanti, l'aumento al 20 per cento della quota europea di consumi derivante da fonti rinnovabili, il *target* obbligatorio del 10 per cento per i biocarburanti usati nel settore dei trasporti, l'aumento del 20 per cento entro il 2020 dell'efficienza energetica a livello europeo e 1'impegno vincolante di ridurre di almeno il 20 per cento in Europa le emissioni di CO2. Ora questo pacchetto di misure dovrà essere contrattato Stato per Stato e la cosa non sarà certamente semplice, ma si tratta comunque di un passo importante perché per la prima volta a livello ufficiale europeo il Governo di centro-destra lo aveva fatto in un Consiglio informale dei ministri dell'energia e dell'ambiente a Montecatini - sono state considerate prioritariamente le convergenze delle politiche ambientali con quelle energetiche nella lotta al mutamento climatico. Gli interventi necessari per centrare gli obiettivi di Kyoto e andare oltre li abbiamo tutti chiari e ci sono strumenti e risorse economiche per avviarli, ma - e di questo sono tutti convinti - la sfida sul clima si gioca prioritariamente a livello politico. I maggiori ostacoli infatti sono rappresentati dalla riluttanza di alcuni Paesi ad impegnarsi e dalle resistenze, sempre minori ad onor del vero, di alcuni settori produttivi. Anche l'industria deve capire definitivamente che Kyoto può rappresentare una grande occasione per rendere concreta la visione dell'ambiente come occasione di sviluppo e di crescita per l'economia. Sembra peraltro che questa visione stia prendendo piede e le parole pronunciate in un'intervista dalla vice presidente di Confindustria, la dottoressa Marcegaglia, vanno in questa direzione. Marcegaglia osserva, infatti, che 1'industria italiana vuole partecipare alla lotta ai cambiamenti climatici che può diventare un'opportunità seria di innovazione tecnologica in cui l'Italia potrebbe avere una *leadership*. Naturalmente - dice la dottoressa Marcegaglia - Governo ed Unione Europea dovranno fare la loro parte convogliando investimenti pubblici sulla ricerca e sull' innovazione, investimenti che possono servire da volano per quelli privati. Per avviare questo percorso, che riesca a far diventare l'ambiente una vera opportunità di sviluppo e vincere la sfida del clima, è necessaria però una politica concreta, pragmatica e non basata soltanto su annunci, una politica che può essere anche *bipartisan*, perché l'ambiente non ha colore politico. Prova di ciò la ricetta fornita nelle settimane scorse dai ministri D'Alema e Bersani, che non è affatto diversa da quella portata avanti nei cinque anni di governo dalla Casa delle Libertà. La nostra mozione per realizzare questa politica ha individuato un cammino in sei tappe, che potrà, da una parte avere, effetti benefici sulla protezione del clima globale e, dall'altra, risolversi in una nuova crescita per l'economia. Tale cammino si può così sintetizzare: in primo luogo, calibrare in maniera corretta il sistema europeo dell'*emission trading* in modo da evitare che settori industriali italiani ad alta efficienza paghino, attraverso l'acquisto di quote, lo sviluppo di settori europei meno efficienti. In secondo luogo, proseguire sulla strada dell'utilizzo dei meccanismi flessibili previsti dal Protocollo di Kyoto. I progetti di cooperazione internazionale già avviati, soprattutto nei settori energetici, forestali ed industriali, potrebbero consentire una riduzione equivalente fino a 60 milioni di tonnellate di anidride carbonica l'anno, con un costo inferiore di oltre il 50 per cento rispetto a quello necessario per i programmi in ambito nazionale, ottenendo così il risultato di promuovere i progetti di imprese italiane a livello internazionale, soprattutto nelle economie emergenti, come dimostra il successo del programma in Cina avviato dal precedente governo. rifinanziare il Fondo istituito presso la Banca mondiale al fine di promuovere i progetti di cooperazione. Questa è un'iniziativa avviata per prima dall'Italia che permette di sviluppare progetti ed acquisire crediti. investire nelle energie rinnovabili e nel risparmio energetico e incentivare le nuove tecnologie energetiche che daranno vantaggi all'ambiente, ma anche alla competitività delle imprese nazionali. In quinto luogo, avviare programmi di adattamento alle conseguenze dei cambiamenti climatici per mitigarne gli effetti. In sesto luogo, scorporare gli investimenti per Kyoto dal Patto di stabilità.

europea, quindi il problema del riscaldamento globale è essenzialmente un problema energetico e rappresenta la più seria minaccia per il futuro dell'umanità e della biodiversità; Se la salvaguardia delle scorte di energia sembra ancora essere l'obiettivo prioritario delle agende politiche internazionali e nazionali, la gravità delle conseguenze legate al cambiamento climatico dovrebbe convincere i Governi a scelte più radicali nel contrastare l'uso di combustibili fossili. Finora sembra che gli unici soggetti preparati ad affrontare il surriscaldamento terrestre siano le grandi compagnie assicurative, le quali devono far fronte all'esponenziale crescita dei danni provocati da fenomeni atmosferici estremi. climatico) ha indicato, senza ombra di dubbio, nell'attività umana la causa dell'aumento delle temperature globali. Quasi il 90 per cento dell'energia mondiale deriva dai combustibili fossili, che per produrla devono essere bruciati generando anidride carbonica nell'atmosfera, uno dei gas maggiormente responsabili dell'effetto serra. Secondo il rapporto presentato dall'IPCC, negli ultimi 200 anni si è registrato un aumento della concentrazione di anidride carbonica nell'atmosfera di oltre il 35 per cento, mentre le temperature terrestri sono salite di circa 0,8 gradi centigradi, rispetto ai livelli preindustriali. Nel nostro Paese, tra l'altro, i cambiamenti climatici si sentono e si sentiranno di più che in altre parti del mondo. Le due regioni del pianeta che risponderanno in maniera più forte all'aumento delle temperature globali sono il Mediterraneo e l'Europa orientale. Ad affermarlo è una ricerca dello scienziato italiano Filippo Giorgi, che fa parte del prestigioso IPCC. Per quanto riguarda l'Italia, all'analisi dell'IPCC vanno aggiunti altri effetti particolarmente allarmanti, quali la progressiva desertificazione e la conseguente mancanza di acqua, dovuta allo spostamento verso Nord dell'anticiclone delle Azzorre, accompagnati da una probabile deforestazione. La crisi idrica del nostro Paese è allarmante e per questo nella mozione chiediamo al Governo di intraprendere politiche forti di riduzione degli sprechi e di favorire la gestione pubblica dell'acqua. A fronte di un aumento medio della temperatura mondiale di 0,65 gradi nell'ultimo secolo, in Europa l'aumento della temperatura è stato, infatti, di 0,95 gradi. In Italia, secondo i dati dell'APAT, in soli 24 anni (dal 1980 al 2004) l'aumento è stato di 1,58 gradi: il doppio della media mondiale secolare. Nella relazione dell'IPCC (che stranamente non è di facile reperibilità in versione integrale, perché - a quanto pare - è stata giudicata troppo catastrofica ed allarmante dai settori industriali), viene inoltre sottolineato il fatto che le capacità naturali di assorbimento stanno diminuendo e sono attualmente in grado di assorbire meno delle metà delle emissioni antropogeniche globali, mentre il resto si accumula in atmosfera e vi permane anche per millenni. Il professor Rubbia, che abbiamo ascoltato in Commissione ambiente nel corso di un'indagine conoscitiva sui cambiamenti climatici, ha precisato, ad esempio, che la metà dell'anidride carbonica sprigionata durante l'incendio di Roma ai tempi di Nerone è tuttora presente nell'atmosfera. Questo implica che la concentrazione di anidride carbonica è proporzionale alla quantità complessiva emessa e non alla intensità o alla velocità di accumulo. Ne consegue quindi che, seppure le misure previste dal Protocollo di Kyoto tese a modificare la velocità di accumulo fossero integralmente applicate, produrrebbero solo un ritardo di appena sette anni nel processo di accumulazione delle emissioni. Misure ben più serie sono quindi necessarie per riuscire a controllare in maniera duratura la concentrazione di anidride carbonica, nel tentativo di limitare l'aumento della temperatura terrestre a più 2 gradi rispetto ai livelli del 1990. È per questi motivi che, a due anni dall'entrata in vigore del Protocollo di Kyoto, l'Unione Europea chiede a gran voce un accordo globale sul cambiamento climatico in grado di succedere al Protocollo nel momento della sua scadenza nel 2012 e di rispondere all'urgenza di procedere a riduzioni più drastiche delle emissioni di gas serra. Sicuramente quello del cambiamento climatico è un problema che che è meglio affrontare a livello internazionale. Tuttavia, questo non vuol dire che possiamo permetterci di attendere che altri Paesi si impegnino prima di intraprendere delle azioni utili a diminuire la nostra dipendenza dall'importazione di combustibili fossili e a colmare il *gap* tecnologico che ci separa da altri Paesi europei. Il ritardo che ci portiamo dietro grazie al precedente Governo è già sufficientemente oneroso e la nostra posizione in Europa e nel mercato globale non può essere ulteriormente aggravata. Aspettare che siano gli Stati Uniti ad agire, o approfittare della titubanza russa come fece il Governo Berlusconi nel corso dei negoziati sul Protocollo di Kyoto nel 2005, affossando di fatto il Protocollo pur di svolgere un ruolo ancillare nei confronti degli Stati Uniti, non è una soluzione. L'unica via intrapresa dal precedente Governo e che l'ex ministro Matteoli intende riproporre oggi nella sua mozione per ridurre le emissioni, è stata quella di comprare crediti di emissione invece che di investire nell'efficienza, nel risparmio e nelle nuove tecnologie pulite. Comprare crediti significa o comprare da chi non è materialmente in grado di inquinare o comprare innovazione e le relative tecnologie da Paesi con elevati livelli di efficienza, assumendo così soltanto i costi degli impegni assunti con Kyoto e non le opportunità. del Protocollo di Kyoto, infatti, è nel senso di intenderlo come una spinta all'investimento nella ricerca e nelle nuove tecnologie pulite, che hanno risvolti importanti su scala mondiale e che permettono notevoli margini di efficienza energetica e di risparmio. Se la comunità umana continua a consumare combustibili fossili per generare energia, oltre ad accrescere le emissioni, accelerando gli effetti negativi del cambiamento climatico, porterà all'esaurimento delle fonti tradizionali di energia. La disponibilità di carbone, petrolio e gas è infatti limitata e secondo alcuni studi si aggirerebbe intorno ai 30-40 anni il termine per l'esaurimento. Questo vuol dire che presto, se non noi, i nostri figli si ritroveranno su un pianeta abitato da quasi dieci miliardi di persone che non avranno accesso ad abbondanti scorte energetiche a basso costo. Tale scarsità delle risorse porterà necessariamente con sé guerra e distruzione. Le possibili soluzioni a questo scenario apocalittico possono essere rintracciate soltanto nel miglioramento dell'efficienza energetica e nello sviluppo delle fonti di energia rinnovabile. Politiche che incoraggiano una produzione e un uso più efficiente dell'energia possono contribuire ad evitare quasi l'80 per cento delle emissioni di anidride carbonica e questo contribuirebbe anche ad una significativa riduzione delle importazioni di gas e petrolio. Inoltre, i costi economici di tali politiche sostenibili sarebbero più che compensati dai benefici connessi ad una maggiore efficienza energetica. Lo stesso Commissario europeo per l'energia ha affermato che «l'efficienza energetica è un elemento cruciale per l'Europa: se agiamo adesso, il costo diretto dei nostri consumi energetici potrebbe ridursi di oltre 100 miliardi di euro l'anno entro il 2020 e ogni anno eviteremo di produrre circa 780 milioni di tonnellate di anidride carbonica». Tra gli obiettivi dell'Unione Europea, finalizzati nel Vertice del 9 marzo scorso, c'è quello di diminuire di un quinto i consumi energetici e di aumentare l'energia prodotta da fonti rinnovabili al 20 Tuttavia, si tratta di obiettivi definiti al ribasso, che potrebbero, e dovrebbero, essere elevati nel caso in cui si impegnassero anche gli altri Paesi industrializzati. È evidente che, a due anni dall'entrata in vigore di Kyoto, gli impegni presi dal nostro Paese con il Protocollo devono essere ripensati anche in funzione dei più stringenti obiettivi fissati di recente dall'Unione Europea per il periodo successivo al 2012. È quello che sta facendo in queste ore il Governo britannico, che propone di abbassare addirittura del 60 per cento le emissioni di gas serra entro il 2050. Certo, occorre vedere con quale *mix* energetico si intende raggiungere un simile abbattimento rifiutando l'utilizzo del nucleare, tuttavia si tratta pur sempre di un'encomiabile iniziativa, che andrebbe seguita dal nostro Governo. L'Italia avrebbe dovuto ridurre le emissioni del 6,5 per cento al 2008-2012 rispetto al 1990, eppure, ad oggi, le emissioni sono aumentate del 13 per cento. Le soluzioni si chiamano fonti rinnovabili, riduzione dei consumi e miglioramento dell'efficienza energetica. esempio è una sorgente di energia assolutamente straordinaria: basti pensare che, per ogni metro quadro di terreno della zona tropicale, potremmo arrivare ad ottenere ogni anno energia corrispondente a 1,5 barili di petrolio. Per rappresentare la quantità di energia che può produrre il sole, che è straordinaria, possiamo immaginare che ogni anno un metro quadro di deserto produca un barile di petrolio. Ad esempio, se l'Arabia Saudita, ossia il Paese che maggiormente abbonda di petrolio, dotasse di adeguati sistemi per la produzione di energia solare una porzione di territorio pari ad un millesimo della propria superficie, produrrebbe una quantità di energia equivalente a tutto il petrolio e il gas naturale che oggi estrae. Quindi, l'Arabia Saudita potrebbe mantenere la sua capacità di produzione energetica rimpiazzando quella di origine fossile con la copertura con specchi solari dell'un per mille della sua superficie. Tra i motivi del ritardo italiano, al primo posto rientrano i perversi incentivi alle fonti cosiddette assimilate, il tanto discusso CIP6 che ancora ieri ha dimostrato quanto siano pesanti e pressanti le azioni delle *lobby* economiche esternamente a questo Palazzo nel continuare a volere questa truffa legalizzata che ha incentivato le fonti assimilate e, soprattutto, il sistema degli inceneritori nel nostro Paese. Per questo chiediamo al Governo di mantenere la promessa fatta in sede di finanziaria e di eliminare gli incentivi perversi alle fonti che rinnovabili non sono. Inoltre, non sembra condivisibile la scelta del Governo di rilanciare il carbone, definito «pulito» per via delle moderne tecnologie che dovrebbero consentire di ridurre le emissioni inquinanti. Certamente, oggi siamo in grado di ridurre significativamente le emissioni di particolato e di altre particelle, ma questo non toglie che bruciando un chilo di carbone si producono 3,5 chili di anidride carbonica. Si tratta di una semplice reazione chimica e non c'è verso di modificarne gli effetti: ogni chilo di carbone bruciato produce 3,5 chili di anidride carbonica a cui va aggiunto un effetto moltiplicativo per 100 di riscaldamento dovuto all'effetto serra già in atto. Anche il beneficio dell'utilizzo di biomasse va comunque messo in relazione all'energia impiegata nei trasporti e all'inquinamento che questi hanno prodotto. La biomassa ha un basso impatto ambientale, ma questo vale soprattutto se si utilizzano scarti di lavorazioni agricole e industriali, legno recuperato o piante coltivate *ad hoc*. Le cose cambiano se il legno proviene da migliaia di chilometri di distanza, da foreste di cui viene intaccata la biodiversità. Il legno che arriva dal Centro e dal Sud America, o spesso dall'Africa, inoltre, ha una filiera difficile da controllare e il rischio di incappare in tagli illegali è concreto. Meglio sarebbe una filiera corta, distretti agroenergetici con un raggio massimo di 50 chilometri. Malgrado l'appurata brevità delle disponibilità di combustibili fossili, ci sono oltre un miliardo di automobili in funzione, che producono ogni anno 4 miliardi di tonnellate di anidride carbonica. Come ha illustrato, con estrema chiarezza, il professor Rubbia ogni automobile in circolazione emette ogni anno una massa di anidride carbonica pari a 4 volte il suo peso. Siccome ogni anno vengono emessi 20 miliardi di tonnellate di anidride carbonica, questo vuol dire che soltanto le automobili contribuiscono per un quinto all'inquinamento mondiale. Se si pensa che in Italia ci sono circa 20 milioni di automobili, vuol dire che esse producono circa 160 tonnellate di anidride carbonica. Questo implica necessariamente il ripensamento di politiche incentivanti per il traffico su gomma, anche per le automobili definite «verdi», «pulite» o «ecologiche». Per questo chiediamo con forza un potenziamento delle infrastrutture di pubblico trasporto, prima di intervenire con grandi opere che spesso di grande hanno soltanto l'immensa inutilità. Con la mozione che presentiamo,

Oggi non siamo molto soddisfatti. Avremmo gradito una discussione più ampia ed articolata, una presenza maggiore di senatori vista anche l'importanza che la Presidenza ha voluto conferire a questa giornata.

la questione del cambiamento climatico ha assunto il carattere di vera e propria urgenza e, soprattutto, è diventata centrale nella discussione internazionale. internazionale. Vi è ormai un consenso ampio da parte di tutta la comunità scientifica internazionale sulla questione del cambiamento climatico.

la stessa Unione europea ha verificato la stretta correlazione tra cambiamento climatico, politiche dell'energia e politiche dei trasporti,

con il recente passato. Ciò deve rappresentare un elemento cardine accanto ad un efficace coordinamento con Regioni ed Enti locali per l'assunzione da parte del nostro Paese delle iniziative, in tutte le sedi internazionali e nell'ambito delle istituzioni comunitarie, per l'attivazione di misure finalizzate alla sostenibilità ambientale e alla lotta al cambiamento climatico.

Oggi, invece, i dati scientifici sono inoppugnabili da questo punto di vista e dimostrano con chiarezza che ciò è strettamente connesso alle attività antropiche e alla crescita delle emissioni di gas serra.

che verrà resa nota per esteso il prossimo 6 aprile a Bruxelles, confermano le valutazioni scientifiche sugli impatti presenti e futuri del mutamento climatico prevedendo un appello ai Governi il mondo per scelte decise ed efficaci sul cambiamento climatico, anche alla luce del fatto che nel maggio prossimo a Bangkok il terzo gruppo di lavoro IPCC presenterà le proprie conclusioni sulle modalità e gli strumenti per affrontare il problema; il Consiglio europeo ha definito, in data 9 marzo 2007, alcuni obiettivi prioritari in materia energetica e ambientale,

un obiettivo vincolante di una quota del 20% di energie rinnovabili sul consumo energetico complessivo dell'Unione europea sempre entro il 2020; Ilnostro Paese purtroppo registra, a causa delle politiche inefficaci ed assolutamente modeste degli anni passati, un ritardo rispetto agli obiettivi previsti dal Protocollo di Kyoto:

di conseguenza della seconda fase che l'Europa vuole portare avanti, è rappresentata dal fatto che gli impegni hanno una veste legale: non sono soltanto impegni politici generici, ma hanno un effetto preciso, puntuale e riscontrabile.

Secondo il Libro bianco sui trasporti della Commissione europea, i trasporti sono tra i maggiori responsabili dell'inquinamento urbano determinando il 40 per cento delle emissioni di CO2.Anche secondo i dati APAT sulla qualità dell'ambiente urbano, presentati recentemente, con riferimento a 24 città capoluogo di Provincia, il trasporto su strada costituisce la principale sorgente emissiva di PM10, benzene, monossido di carbonio, ossido

e la ricerca in campo energetico. Ciò deve passare attraverso un'iniziativa volta non solo a rafforzare la cooperazione internazionale già in sede di G8 Ambiente (che avrà luogo tra qualche giorno), ma anche in sede di coinvolgimento degli enti locali, di responsabilizzazione del mondo delle imprese per ridurre le emissioni, a partire dall'attuazione di efficaci piani nazionali di allocazione delle quote di emissione, in modo da premiare le iniziative più innovative nel campo della produzione, della distribuzione e del consumo di energia evidente, però, che il vigente meccanismo del mercato dei titoli di emissione determina il trasferimento di risorse da interventi concreti a interventi poco monitorabili e di scarso impatto sulla vita concreta delle popolazioni. Questo Governo e questa maggioranza già con la legge finanziaria per il 2007 - lo vorrei ricordare perché stiamo cominciando ad avviare politiche in controtendenza rispetto al passato per far fronte rapidamente

da garantire un'inversione di tendenza e, soprattutto, un forte impegno sul fotovoltaico, sul solare e sulla ricerca applicata alle energie rinnovabili e sullo sviluppo delle agroenergie incentrato su politiche di filiera corta e sul protagonismo diretto degli imprenditori agricoli. legge finanziaria, sono stati approvati rilevanti interventi volti a rafforzare il tema strategico dell'efficienza e del risparmio energetico. È stato istituito un fondo rotativo per il finanziamento delle misure finalizzate all'attuazione del Protocollo di Kyoto. Si comincia finalmente ad applicare il sistema di incentivazione delle fonti rinnovabili che discende dalla direttiva CE n. 77 del 2001 e che ha ricevuto

adeguata per contrastare i cambiamenti climatici, occorre che l'insieme delle questioni ambientali sia posto al centro dell'azione di Governo, come si sta già cominciando a fare. Infatti, il recupero di una

infrastrutture, torno a sottolinearlo, riveste un'importanza strategica per uno sviluppo sostenibile del Paese. È stato dato avvio, altresì, alla riqualificazione delle politiche e degli investimenti pubblici

deve essere sempre più indirizzata verso politiche di risparmio mirate nei settori in cui si registrano ancora ampi margini di spreco o di dispersione, senza che tale risorsa sia assoggettata solo alle logiche del profitto. Una seria politica dell'acqua, infatti, è strettamente correlata ad una politica

e misure ancora più incisive da attivare non solo in ambito internazionale, ma anche ovviamente e principalmente nel nostro Paese. È necessario poi avviare, in sede comunitaria, sia una riflessione sull'incisività del meccanismo della compravendita di titoli di emissioni emissioni sia adeguate iniziative volte alla nascita di un mercato interno di titoli di emissione che sia davvero efficace, monitorabile e concreto, anche attraverso forme di controllo sull'origine delle emissioni stesse, verificando altresì quali tra i comparti a alto impatto ambientale debbano, essere attenzionati. Bisogna predisporre, un piano energetico che abbia l'obiettivo di superare la dipendenza dai combustibili fossili; avviare politiche serie per uscire dall'era del petrolio - questa è la nuova emergenza mondiale - e favorire il risparmio e l'efficienza energetica.

definire una revisione dei meccanismi di incentivazione delle fonti rinnovabili che consenta anche lo sviluppo della filiera del legno, dei residui agricoli, del biogas, dell' olio vegetale, sostenendo impianti di piccola e media dimensione, fortemente integrati con i distretti energetici locali e gestiti dagli agricoltori. Occorre il metodo della trasparenza e della pianificazione anche nella gestione del territorio, promuovendo un maggiore impegno per affrontare il dissesto idrogeologico e rafforzare la difesa del suolo; favorire il rilancio del sistema dei parchi e delle aree protette nazionali; definire una strategia nazionale, in attuazione della Convenzione internazionale sulla biodiversità; rafforzare un programma d'intervento sulle grandi aree urbane che rappresentano oggi una grande emergenza e su cui è possibile

crescita attenta e sostenibile che può produrre effetti per l'ammodernamento del nostro sistema produttivo, per la salvaguardia del nostro Paese e per l'occupazione.

che, di norma, ci si iscriva il giorno prima. Ebbene, ormai ci siamo abituati al fatto che questa regola non viene più rispettata: vorrei capire, se non viene rispettata abitualmente, se non viene rispettata secondo i giorni, se non viene rispettata secondo chi presiede, se non viene rispettata secondo l'argomento. In tal modo, infatti, potremmo disciplinare i nostri lavori, nel senso che se sappiamo che non viene rispettata mai, ci abituiamo; se invece non viene rispettata a fasi alterne, ci informeremo di volta in volta, presso gli Uffici, su quali regole si intende applicare. penso che una volta per sempre la Giunta per il Regolamento debba decidere come si applica il Regolamento, in maniera tale che noi lo rispettiamo e sappiamo come dobbiamo comportarci. Altra questione, ieri il collega Manzione ha sollevato una serie di questioni sulle trasgressioni permanenti del Regolamento e, in particolare, ne ha segnalate due. poco dopo l'intervento del collega Manzione, vi è stata l'ennesima trasgressione: il Presidente di turno dell'Assemblea,

che viene approvato; dopodiché, se vi è la possibilità che il calendario venga modificato, dobbiamo adeguare la nostra informazione a tale eventualità.

si prevede che nella Conferenza dei Capigruppo di martedì mattina vi sia la possibilità, in contrasto con il Regolamento, di modificare il calendario. Se mi dà lumi su questi punti,

Lei dice che ieri, in sede di votazione, il senatore Manzione ha fatto dei rilievi sulle trasgressioni al Regolamento; leggerò le osservazioni del senatore Manzione, che meritano l'attenzione dovuta. Per quanto riguarda poi il tempo della votazione, io ho la più assoluta fiducia nel senso di responsabilità e nelle capacità dei Vice presidenti che si alternano alla Presidenza dell'Assemblea, cui è riconosciuta questa capacità da parte di tutti. Quindi, non riesco a capire quali valutazioni ci siano state

Il Regolamento parla chiaro: in caso di unanimità, il calendario resta così stabilito, in caso di disaccordo, stabilisce l'Aula. Non riesco a capire lo spirito e neanche la *ratio* dell'intervento del collega Boccia. Credo che questo sia un punto fermo dal quale non si possa derogare, poi è tradizione che i senatori che svolgono

sono volti ad incentivare fonti energetiche rinnovabili comprendendo le fonti assimilabili. I ministri Bersani e Ronchi, Governi successivi, decisero di estendere l'utilizzo delle risorse riservate alle fonti di energia rinnovabile agli impianti di trattamento dei rifiuti. Questa è la storia dei CIP6.

Sodano. Perché io sarei legato alle *lobby*? Perché faccio riferimento anche a questi sei impianti, che hanno svolto le gare d'appalto quando c'era il CIP6, hanno ottenuto finanziamenti - perché la realizzazione di questi impianti

riportiamo la discussione nei termini giusti: c'è una divergenza, ma non accuso il collega Sodano di essere legato alla *lobby* di chi ha già gli impianti. Pregherei il senatore Sodano di non dire che l'ex ministro e senatore Matteoli è legato alla *lobby* di quei quattro imprenditori, perché non è così. La mia posizione è nella logica e soprattutto nel buonsenso. Detto questo, c'è un altro aspetto che vorrei sottolineare (lo farà meglio di me dopo il senatore Battaglia, così come prima di me lo ha fatto il senatore Mugnai). La mozione presentata

per la sensibilità dimostrata nei giorni scorsi nel disporre il dibattito di questa mattina e per la risposta che ha dato al collega Boccia, per ampliare al massimo il dibattito su un argomento così importante come l'ambiente

indubbiamente la questione all'esame oggi, fortunatamente, non è più, nella consapevolezza di molti senatori e di una rilevante e crescente parte dell'opinione pubblica, pubblica, un problema riservato alla meritoria battaglia del partito dei Verdi o alle sensibilità ambientali del Paese.

e prendo atto con piacere che persino dal centro-destra, che irrideva il ruolo delle tematica ambientale nonché il Protocollo di Kyoto, vi sia invece la presa d'atto che la questione esiste, eccome. Credo, quindi,che vada dato atto al Governo, per la parte relativa alla nuova edilizia, di aver fatto dei passi avanti Pecoraro Scanio di essersi battuto e di aver ottenuto dei risultati, ma che insieme si debba convenire con quanto detto dal senatore Sodano e cioè che bisogna camminare più speditamente e in modo più stringente. Dico in modo più stringente perché la contraddizione è lampante anche nel comportamento sul territorio: mi riferisco alle questioni che

non sia navigabile e sappiamo che la prospettiva è largamente peggiore. Quindi, coerenza tra scelte e problematiche che si affrontano in sede legislativa e comportamento sul territorio: visto che le risorse sono scarse, è indubbio che sprecarle è un errore. Credo anche che, dal punto di vista del suolo e dei piani urbanistici, occorra agire con lungimiranza - uscendo dallo scadimento della nuova generazione degli amministratori, che puntano ad arrivare a fine mandato e poi si arrangerà chi verrà dopo - nell'edilizia che riguarda gran parte dei litorali italiani. Sappiamo tutti che il relatore europeo sui temi dell'ambiente lui è dei Paesi Bassi, dove forse il problema è più cogente) ha detto che ora abita a 150 chilometri dal mare e suo nipote abiterà nella stessa casa a 75 chilometri dal mare; quindi,i piani urbanistici e l'uso del territorio

si stabilisse un percorso virtuoso, in base al quale un cuneo anche di maggior sconto fosse applicato a quelle aziende che si fossero impegnate ad introdurre innovazioni di processo o di prodotto per quanto riguarda l'impatto ambientale ed il consumo energetico, perché è tutta una politica che va ripensata e credo che la sinistra debba camminare più rapidamente su questi temi. temi. Affronterò questa discussione partendo da una posizione di difetto rispetto ai colleghi della sinistra, perché culturalmente ed ideologicamente non sono nemmeno chiuso al tema del nucleare, quindi riceverò molte critiche, ma credo che finché

non ci si debba chiudere rispetto a quest'elemento che determina una prospettiva complessiva per l'umanità. È sicuramente interessante anche la cultura del regresso dello sviluppo (anche se il termine corrente è diverso), che Grillo ed altri ambientalisti sostengono, ma credo che nemmeno una dittatura potrà imporre al nostro Paese o ad altri un arretramento di gran parte degli stili e dei consumi di vita, pur essendo una battaglia che va culturalmente fatta.

la storia del movimento operaio ha portato alla pubblicizzazione, lo stesso articolo 43 della nostra Costituzione parla di pubblicizzazione dei servizi di pubblica utilità nel nostro Paese. Do atto al partito

nel momento in cui il progresso scientifico va rapidamente collegato ai processi produttivi ed alle modalità di vita dei cittadini, nel momento in cui il trasporto incide, nel momento in cui il tema energetico è quello su cui si fanno le guerre e che determina il futuro di gran parte dell'umanità,

Applaudo e accolgo con favore la proposta presente nelle mozioni dell'Unione relativa all'indizione della Conferenza nazionale sull'acqua. Lo sforzo da sostenere è grande. Molto compete a questa sede legislativa, ma ci sono un dibattito culturale, una mobilitazione, un coinvolgimento dei cittadini sulla gravità del problema, rispetto al quale tutti siamo purtroppo inadeguati.

premetto subito di essere pienamente a favore della mozione che ha come primo firmatario il presidente Matteoli, nei confronti della quale vorrei fare alcune considerazioni, riferite in particolare a tre suoi punti. Inizio con alcune considerazioni di carattere generale. Sul nostro pianeta è in atto un cambiamento climatico caratterizzato dal progressivo innalzamento delle temperature dell'atmosfera; in termini di temperatura media al suolo, con tutti i limiti che questo concetto di temperatura media presenta e sono gravi, tale innalzamento è stato nel secolo scorso di circa 0,6 gradi, di cui 0,4 gradi avvenuti negli ultimi quattro decenni. Cambiamenti climatici di questo tipo non sono assolutamente eccezionali nella storia del nostro pianeta. Senza scomodare fenomeni imponenti e ricorrenti come le grandi glaciazioni, considerando anche solo gli ultimi mille anni della nostra storia, si sono avute nei primi tre-quattro secoli temperature più alte di quelle attuali attuali (queste temperature hanno consentito - ad esempio - una temporanea occupazione della Groenlandia da parte dei Vichinghi, da cui il nome della fredda isola, nonché la coltivazione della vite in Gran Bretagna). Successivamente, in particolare a partire dal 1650, vi è stato un cospicuo raffreddamento del clima fino a tutto il secolo XIX (tanto che per questo periodo gli scienziati parlano di piccola glaciazione). Gli scienziati hanno avanzato varie ipotesi circa le possibili cause di queste instabilità climatiche quali: variazioni della concentrazione di gas serra nell'atmosfera (in particolare anidride carbonica);

variazioni del moto della terra attorno al sole; variazioni dell'attività vulcanica; variazioni del coefficiente di riflessione della radiazione solare delle terre emerse (importanti quest'ultime a seguito dell'agricoltura diffusa in tutto il pianeta); variazioni delle correnti oceaniche; impatto di asteroidi; variazioni del contenuto di aerosol nell'atmosfera, e via Per quanto riguarda il riscaldamento globale in atto, la maggioranza degli scienziati ritiene che la causa sia da attribuire all'effetto serra generato dall'anidride carbonica immessa nell'atmosfera per opera dell'uomo mediante la combustione di carbone, petrolio e metano, immissione iniziata circa la metà del secolo XVIII e proseguita fine ai nostri giorni con flussi sempre crescenti. Tuttavia, una parte consistente degli scienziati, e tra questi anche scienziati di grande peso (due nomi tra tutti: quello del professore Fred Singer della Virginia University e del professore Richard Lindzen del MIT di Boston), ritiene che l'attribuzione della causa del riscaldamento globale in atto all'anidride carbonica antropogenica non sia affatto sufficientemente provata. La percentuale di anidride carbonica nell'atmosfera è aumentata dal 1750 ad oggi da circa 280 parti per milione a circa 380 parti per milione, con un aumento del 35 per cento. L'aumento complessivo della quantità di anidride carbonica contenuta nell'atmosfera così avvenuto corrisponde a circa la metà della quantità di anidride carbonica immessa nell'atmosfera dall'uomo mediante la combustione dei combustibili fossili. Attualmente, il ritmo annuale di incremento della percentuale di anidride carbonica nell'atmosfera è in media di circa 1,8 parti per milione. Secondo l'Agenzia Internazionale dell'Energia, nel corso del 2004 nel mondo sono stati immessi nell'atmosfera oltre 26,5 miliardi di tonnellate di anidride carbonica,

cioè 21 anni prima, le immissioni sono state pari a 15,6 miliardi di tonnellate; dunque, sono in crescita. Le immissioni dovute all'Italia nel 2004 sono state pari a 462 milioni di tonnellate, cioè l'1,7 per cento Nell'atmosfera hanno luogo vari effetti serra. Quello di gran lunga principale è dovuto al vapor acqueo che ha percentuali di concentrazione nell'atmosfera molto superiori a quelle dell'anidride carbonica. Oltre all'effetto serra dell'anidride carbonica va tenuto in conto anche quello del metano che, però, attualmente è assai meno importante.

l'anidride carbonica ha ormai prodotto i tre quarti dell'effetto riscaldante dell'atmosfera che si verificherebbe con un raddoppio della concentrazione esistente nel 1750,

che ha avuto un grande sviluppo a partire dal 1970 per effetto delle osservazioni satellitari. È diventata una scienza interpretativa e predittiva solo negli ultimi decenni per merito della disponibilità di supercalcolatori sempre più potenti. Con essi è stato affrontato il compito immane di riprodurre la dinamica straordinariamente complessa delle temperature dell'atmosfera determinata dalle interazioni energetiche e fluidomeccaniche dell'atmosfera, degli oceani e delle terre emerse sottoposte alla radiazione solare e agli effetti dei moti della terra. In tale sistema le variazioni di temperatura dell'atmosfera determinano potenti meccanismi sia di retroazione positiva (tendenti, cioè, a rafforzare le variazioni di temperatura), sia di retroazione negativa (tendenti, cioè, a contrastare le variazioni di temperatura). I codici di calcolo utilizzati attualmente per le previsioni climatiche sono di incredibile complessità. Vi vengono simulate numericamente le moltissime equazioni relative a centinaia di fenomeni di fluidodinamica, di idrodinamica, di scambio termico, di cambiamento di stato (da liquido, a vapore, a stato solido e viceversa), di reazioni chimiche, eccetera. Alcuni di questi fenomeni, come, ad esempio, la dinamica della formazione delle nubi (un fenomeno fondamentale) non sono ancora conosciuti a sufficienza. Per superare le difficoltà dovute a tali incertezze, nei suddetti codici di calcolo un certo numero di parametri sono aggiustati *ex post* utilizzando le serie storiche dei dati disponibili (in particolare, di temperatura). Tali serie storiche, tuttavia, hanno una limitata estensione nel tempo (pochi decenni). Un problema molto serio per questi codici di calcolo, poi, è quello della validazione. Per queste ragioni le previsioni degli aumenti di temperatura dell'atmosfera al 2100, effettuate attualmente anche dai più accurati codici di calcolo climatologico, rischiano di essere affette da rilevanti errori che purtroppo, allo stato, non sono ben valutabili. Un indizio di tale incertezza è segnalato dalla grave discordanza delle previsioni fatte dai diversi codici di calcolo circa l'aumento della temperatura media che dovrebbe verificarsi nel 2100. La disponibilità di grandi quantità di energia a prezzi ragionevoli è assolutamente essenziale per il buon funzionamento delle moderne società industriali e post- industriali quale quella del nostro Paese.

Le altre fonti energetiche sono state: l'energia nucleare (poco più del 6 per cento), l'energia idroelettrica (poco più del 2 per cento) e la combustione di biomasse e rifiuti (poco più del 10 Il contributo di tutte le altre fonti energetiche, ivi comprese tutte le fonti energetiche rinnovabili, non è arrivato all'1 per cento. Con il rapido sviluppo in corso di grandi Paesi come la Cina, l'India, l'Indonesia, il Brasile ed il Sudafrica, la domanda di energia mondiale tende a crescere rapidamente e secondo le previsioni dell'Agenzia internazionale dell'energia il consumo mondiale di energia nel 2030 sarà del 55 per cento superiore a quello attuale. Una frazione importante delle fonti energetiche primarie viene utilizzata per la produzione di energia elettrica; gli impianti necessari per tale produzione richiedono in generale imponenti investimenti (in particolare per gli impianti nucleari e per quelli idroelettrici), inevitabilmente da ammortizzare in decine e decine d'anni. Anche solo per questo si comprende come i sistemi energetici abbiano necessariamente ritmi di evoluzione piuttosto lenti. Se è corretta l'attribuzione del riscaldamento globale in atto all'anidride carbonica presente nell'atmosfera, data la grande inerzia dei sistemi energetici, data l'enorme prevalenza di combustibili fossili nell'approvvigionamento energetico mondiale (come sappiamo oltre l'80 per cento), data la sicura crescita negli anni futuri del fabbisogno energetico mondiale, dato il costo elevatissimo delle fonti energetiche rinnovabili, principale sostituto dei combustibili fossili, la concentrazione dell'anidride carbonica nell'atmosfera nei prossimi decenni non potrà che aumentare. Gli esperti prevedono il raggiungimento di 450-500 parti per milione entro il 2030. Di conseguenza, aumenteranno gli effetti sul riscaldamento globale. Per limitare i danni dovuti a questo riscaldamento (peraltro esagerati nel rapporto di Nicholas Stern) non resta che sviluppare iniziativa di adattamento. Se, invece, il riscaldamento globale in atto non è dovuto all'aumento di concentrazione dell'anidride carbonica nell'atmosfera, ma ad altre cause, come alcuni, pochi, scienziati si ostinano a ritenere, le iniziative di adattamento diventano l'unica mitigazione possibile degli effetti del riscaldamento globale. In parallelo alle azioni di promozione delle fonti rinnovabili, del risparmio energetico, della efficientizzazione degli usi finali di energia, in sostanza in parallelo a tutto questo sforzo di riorientamento dei sistemi energetici (che inevitabilmente prenderà molto tempo data la grande inerzia di tali sistemi) occorre perciò, in ogni caso, intraprendere concrete azioni di adattamento al cambiamento climatico. Non abbiamo alternative. Comunque vadano le cose la «*low carbon economy»*, grande obiettivo del presidente Barroso, non potrà affermarsi a livello mondiale prima di parecchi decenni e ulteriori decenni saranno necessari perché si possano evidenziare i suoi effetti sulla concentrazione di anidride carbonica nell'atmosfera. Dobbiamo perciò deciderci ad eliminare il tabù che finora ha circondato l'obiettivo dell'adattamento, impedendo persino che se ne parlasse.

un'iniziativa altamente apprezzabile, in particolare per il suo principio ispiratore, vale a dire la volontà di assumere una responsabilità collettiva di gestione delle attività umane suscettibili di apportare modifiche importanti all'ambiente terrestre, assunzione da porre in essere tramite accordi sottoscritti da tutti i Paesi del mondo.

utilizzato in ambito europeo con meccanismi particolari. Uno di questi meccanismi è la sanzione di circa 100 euro a tonnellata di anidride carbonica per eventuali esuberi rispetto ai limiti

Le regole stabilite concretamente dalla Commissione europea per l'*European trading system* penalizzano cospicuamente l'Italia: il cittadino italiano ha diritto *pro-capite* di immettere nell'atmosfera anidride carbonica in quantità molto inferiore a quella del cittadino tedesco (poco più della metà) a quella del cittadino tedesco (poco più della metà) e in quantità appena superiore a quella del cittadino francese, ma la Francia, per via del massiccio ricorso al nucleare, produce la propria energia elettrica praticamente senza utilizzare combustibili fossili. Per centrare gli obiettivi stabiliti dal Protocollo di Kyoto, il nostro Paese dovrebbe ridurre - come è già stato ricordato - entro il 2012 la quantità di immissione di anidride carbonica nell'atmosfera del 17-18 per cento rispetto al valore attuale, un valore impossibile da raggiungere. Dovremo, quindi, avvalerci dei meccanismi sussidiari previsti dal Protocollo ed, in primo luogo, dell'acquisto di diritti di emissione nel quadro del mercato ETS, con esborsi che si prevedono cospicui: se il prezzo dei diritti di immissione sarà di 20 euro la tonnellata di anidride carbonica e l'Italia avrà nel 2012 una sovraimmissione di circa 100 milioni di tonnellate di anidride carbonica annui - come molti prevedono - l'esborso sarà di 2 miliardi di euro di euro l'anno, che graveranno sulla già carissima bolletta elettrica dei cittadini italiani. Per ovviare a queste anomalie

questi elementi presso la Commissione europea. In particolare, va ridefinito il meccanismo dell'ETS affinché si abbiano diritti di immissione di anidride carbonica nell'atmosfera più equamente distribuiti tra i vari Paesi membri rispetto a come sono attualmente disposti. In ultimo, segnalo un punto particolarmente importante della mozione 1-00070, là dove impegna il Governo a promuovere nel nostro Paese la produzione di energia elettrica mediante impianti termovalorizzatori dei rifiuti (in particolare, di quelli solidi urbani); questa importante fonte energetica, ingiustamente da noi molto trascurata, è da considerarsi anche in parte una fonte energetica rinnovabile, perché una frazione consistente - tipicamente la metà - dei rifiuti solidi urbani termovalorizzati sono biomasse. *(Applausi

Signor Presidente, nella tornata di ieri un collega, pur partecipando con foga al dibattito sulla risoluzione europea, ne revocava in dubbio l'utilità, dichiarandone la strumentalità ai fini di «perdere tempo», non avendo altro da proporre all'Assemblea. Mi sono convinto, invece, che (sia pure introdotti nel calendario con qualche attenzione) dibattiti come quello di ieri o quello di oggi possono contribuire in modo efficace alla promozione di idee forti e allo stimolo di responsabilità politiche, civili e culturali per l'intero Paese. La sensibilità in tema ambientale non è nuova né opzionale. La mozione 1-00070, a prima firma del collega Matteoli, è un esempio di come anche le politiche ambientali siano confrontabili da fronti politici diversi, pur partendo da talune definizioni comuni di obiettivi praticabili. In essa ho apprezzato soprattutto il realismo con il quale affronta il delicato tema dei rapporti internazionali e delle esigenze di una regia europea nei confronti delle possibili iniziative di collaborazione, soprattutto con le nuovi grandi ed imprevedibili potenze industriali dell'Oriente. La mozione 1-00065, a prima firma del collega Ferrante (che pure io ho sottoscritto), ha optato per centrare soprattutto il tema dei consumi di energia elettrica, sia con riferimento agli obiettivi del Protocollo di Kyoto, sia in considerazione della completa liberalizzazione del mercato elettrico a partire dal 1° luglio prossimo. Si chiede al Governo di muovere leve plurime, con molto pragmatismo, al fine soprattutto di coinvolgere l'utente - cioè il cittadino - in comportamenti positivi, virtuosi. Non sfugge a nessuno l'enorme risvolto economico di ogni scelta in campo energetico; forse qualche ipocrisia in meno rispetto agli interessi privati e pubblici in gioco favorirebbe una maggiore assunzione di responsabilità imprenditoriali e politiche.

Dovremmo cercare di individuare una ripartizione equa, tra minori guadagni per pochi e maggiori risparmi per il maggiore numero di concittadini. E anche un più evidente rigore nei consumi energetici da parte degli enti pubblici (Stato, Regioni, Province e Comuni anzitutto): lo spreco si annida nel riscaldamento, nel raffrescamento e nell'utilizzo indiscriminato e smodato di mezzi di trasporto individuali. C'è un problema culturale di fondo, una condivisione di scelte anche personali, prepolitiche, che deve essere messa in gioco. Se è vero, come ci ricordava il professor Rubbia recentemente in un'audizione presso la 13a Commissione, che la ripercussione dei comportamenti personali e collettivi produce effetti nel medio-lungo periodo, oggi soggiacciamo alle scelte degli anni passati e condizioniamo già le qualità della vita futura dei nostri figli con i nostri attuali comportamenti. Da qui la necessità di diffusi momenti di formazione e anche di scelte di politica economica ambientalmente responsabili (compatibili, come da gergo). L'auspicio è che il Governo raccolga positivamente tutte le sollecitazioni, anche quelle puntuali, emergenti dal dibattito e - forte anche di un programma già particolarmente significativo al riguardo - proceda con determinazione nel perseguimento degli obiettivi di Kyoto e oltre. Un'ultima considerazione mi pare necessaria: nel rapporto tra lo Stato e i Comuni anche la materia ambientale può prestarsi a gestioni non razionali. Credo che lo Stato dovrebbe manifestare, assieme alla capacità d'indirizzo e a quella di controllo (con conseguente sanzione, se necessario), anche una maggiore attitudine sussidiaria, sia attraverso il finanziamento di ogni possibile iniziativa di razionalizzazione e risparmio dei consumi energetici (penso ai piani per il fotovoltaico negli edifici pubblici o alle determinazioni per l'incentivazione e la diffusione dell'uso del metano per autotrazione), sia attraverso premialità consistenti, sempre in termini di finanza pubblica, per risultati particolari o innovazioni significative. I Comuni sono gli enti pubblici più vicini alle cittadine e ai cittadini. Una pianificazione di interventi nella complessa materia della tutela ambientale non può che rimetterli al primo posto, certamente in termini di responsabilità, ma anzitutto in termini di promozione di comportamenti attivi e positivi (e di fiducia:

Non è pensabile che il bene dell'ambiente possa rientrare nell'esclusività di qualcuno o di un parte politica; si ritiene che l'ambiente sia sia quel bene che tutti insieme rincorriamo e tutti insieme vogliamo tutelare, così come ognuno di noi intende tutelare la propria salute

Certamente, non ci possiamo dividere sull'ipotesi della raccolta differenziata che vedrebbe risolto il problema dei rifiuti, tranne che in Campania,

Ci andrei molto piano anche per quanto riguarda le responsabilità contabili, nel momento in cui si ritiene, di fronte a un diritto quesito, quale quello del CIP6, di tornare indietro, creando un danno all'economia di questo Paese.

esperti», «Terra a rischio» sono alcuni dei titoli apparsi sui quotidiani di questi giorni che dimostrano come la consapevolezza dell'emergenza climatica sia ormai entrata a far parte del nostro vivere quotidiano. D'altra parte, proprio negli ultimi mesi, dal mondo della scienza è stata sottolineata, quasi all'unanimità, la responsabilità dell'uomo nella variazione del clima e pochi sono ancora convinti e pochi sono ancora convinti che l'effetto serra non sia imputabile all'uomo. Secondo i rapporti internazionali le emissioni di carbonio, derivanti dall'utilizzo di combustibili fossili, continuano a crescere. Dall'inizio della Rivoluzione industriale di fine '800, quando l'uomo ha iniziato a bruciare grandi quantità di combustibili fossili per produrre energia, il totale annuo di emissioni ha continuato a crescere a ritmo sempre più rapido. Dal 1900 si è moltiplicato per 15 e ogni anno è aumentato del 3 per cento rispetto Il problema del mutamento climatico, come sottolineato in un recente libro dal titolo «Clima: istruzioni per l'uso», di Ferrara e Farruggia, sta proprio nell'ampiezza del mutamento e nella sua scelta temporale. Il clima, infatti, sta cambiando in maniera troppo intensa perché questo non comporti effetti sulle comunità umane, e troppo velocemente È vero che uomo e sistemi naturali hanno saputo sempre adattarsi nei secoli ai cambiamenti del clima, ma si trattava di cambiamenti lenti. Oggi non è più così: se si perturba l'equilibrio del sistema climatico in maniera così massiva, nessuno sa esattamente come e con che velocità potrebbero evolvere le cose. Mancano le certezze assolute, ma il rischio di un significativo cambiamento climatico nei prossimi decenni o entro la fine del 2100 esiste concretamente. Di fronte a questi scenari sempre più preoccupanti, la politica ha cominciato a dare risposte, anche se ancora timide e a volte ambigue. Ma il dibattito che stiamo svolgendo oggi in quest'Aula dimostra con chiarezza che i problemi ambientali attraversano trasversalmente tutti gli schieramenti, proprio perché è in gioco la salute del pianeta e delle generazioni future, nonché l'assetto sociale ed economico della nostra società. Ormai siamo infatti tutti convinti della relazione inestricabile tra salvaguardia ambientale e sviluppo economico. L'economista inglese Nicholas Stern ci ha detto chiaramente che bloccare il cambiamento climatico in atto costerebbe oggi l'1 per cento del PIL mondiale, mentre, se non si prendessero misure, l'economia questo secolo, di avere perdite fino al 20 per cento del PIL a causa dei mutamenti climatici. L'industria sta man mano prendendo contezza che l'ambiente può diventare l'opportunità di sviluppo e che investire in tecnologie amiche del clima può rendere più competitivi sui mercati mondiali. L'Italia, come ha detto un esponente di Confindustria, in questo campo può far scuola e i cambiamenti climatici possono essere il *driver* importante di innovazione tecnologica. Il precedente Governo, e in particolare il Ministero dell'ambiente, proprio per disseminare le tecnologie italiane, aveva avviato numerosi progetti di cooperazione ambientale con i Paesi emergenti che nei prossimi anni saranno i maggiori emettitori di gas ad effetto serra. La eco-cooperazione di maggior successo - come è stato riconosciuto anche in un editoriale del quotidiano «La Stampa» - è stata quella in Cina, dove si sono avviati una serie di progetti di collaborazione (riguardanti bioenergie, energie rinnovabili, trasporti puliti, disinquinamento e altro ancora) che permetteranno alle aziende italiane di entrare nel mercato cinese e, nello stesso tempo, di esportare in quel Paese tecnologie pulite. Per la salvaguardia del clima, come sono ormai tutti convinti, serve infatti un approccio globale. Le riduzioni di gas serra producono i suoi effetti sul clima ovunque avvengono e, per un Paese come l'Italia, in cui il sistema produttivo gode di un'alta efficienza energetica, la possibilità la possibilità di avviare progetti di riduzione delle emissioni in Paesi emergenti serve sia alla competitività del Paese, sia nei confronti dello Stato. Secondo calcoli fatti, se l'Italia, per rispettare il Protocollo di Kyoto, dovesse intervenire per ridurre le emissioni soltanto all'interno del proprio sistema produttivo, avrebbe costi tre o quattro volte superiori a quelli della Germania e degli altri Paesi dell'Unione europea, meno efficienti a livello energetico. Tenendo conto di questi dati, l'Italia (che, tra l'altro, come riportato dall'Agenzia europea dell'ambiente, ha tra le più basse emissioni di CO2 *pro capite*) dovrebbe focalizzare il suo intervento, non solo all'interno del suo sistema energetico produttivo (dove rischia però di raschiare il fondo del barile), ma anche, come ha fatto il precedente Governo, nei Paesi extraeuropei. Paesi extraeuropei. In questo modo, se il nostro fine è la lotta ai cambiamenti climatici e non la difesa di posizioni ideologiche, un provvedimento per la riduzione delle emissioni di gas serra dovrebbe prevedere interventi sostanziosi in Paesi come l'India, la Cina e così via.

Signor Presidente, colleghe e colleghi, credo sia fuori discussione che negli ultimi mesi, nell'ultimo anno, l'allarme ambientale, in particolare sul clima, è tornato prepotentemente nel dibattito, anche politico. Naturalmente per noi ambientaliste è un problema molto molto noto, con anche molte incertezze e molte scelte che sono state fatte in passato che hanno dato anche risultati apprezzabili. Ma resta una questione di fondo sulla crescita e sullo sviluppo economico che è insostenibile su scala planetaria. II problema essenziale che abbiamo di fronte, come Paese occidentale,

i germi del fallimento su scala planetaria; non è estensibile a tutti, altrimenti arriveremmo rapidissimamente, molto più rapidamente di quello che immaginiamo, al collasso.

però ricordare che sul tema ci sono ormai numeri, tendenze e studi riconosciuti, in modo direi universale dal mondo scientifico, pur naturalmente con qualche eccezione, di cui il rapporto dell'IPCC, presentato a Parigi nel febbraio 2006, è sicuramente un autorevole riconoscimento e ci esorta a molte azioni per cambiare rotta e a farlo anche in fretta, perché gli effetti a cascata di queste misure sono indispensabili. Voglio anche ricordare che quello ambientale non è solo un problema di benessere per noi noi cittadini del mondo occidentale, ma è un problema di sopravvivenza per molte parti del pianeta. Voglio ricordare che ben 2 miliardi di cittadini del mondo sono esposti a desertificazione ed aridità, cioè a fenomeni di degrado del territorio tali da minacciare la loro stessa sopravvivenza e il loro diritto di sussistenza. Questo è anche il problema ambientale. Allo stesso modo, certo, lo riconosciamo ed è indiscutibile, i consumi crescenti, che generano certamente benessere, lo fanno però in modo altamente diseguale nelle diverse parti del pianeta.

Voglio usare un fatto di cronaca, sicuramente positivo, la liberazione dei due lavoratori dell'ENI che erano stati rapiti nel Delta del Niger,

se non altro, dalle immagini televisive che facevano vedere queste piattaforme petrolifere sul Delta del Niger, questo straordinario ecosistema, con accanto dei villaggi di popolazioni residenti, alla fame, senza lavoro, senza sanità, senza scuola. Credo allora che al Governo vada anche chiesta un'azione, perché, ovviamente insieme allo sviluppo industriale e al recupero di risorse, sicuramente utili al mondo occidentale, vi siano anche degli obblighi di occupazione, di servizi, di dialogo con le popolazioni locali che non possono essere semplicemente rapinate in nome di un diritto internazionale. C'è anche un altro aspetto che voglio ricordare, è un tema molto delicato ma lo voglio affrontare ugualmente, quello della crescita della popolazione. Noi oggi siamo 6 miliardi, nel 1960 eravamo 3 miliardi, gli studiosi dicono che nel 2050, fatte salve tendenze che naturalmente possono essere corrette in ogni direzione (sono dati tendenziali), saremo 9 miliardi. È evidente che la crescita della popolazione, dovuta sicuramente anche al benessere, alla consapevolezza, al progresso scientifico, che tutti naturalmente apprezziamo, ha però dei limiti di capacità di carico di questo pianeta che non possiamo eludere e sui quali dobbiamo riflettere. Naturalmente, le scelte individuali vanno sempre promosse e rispettate ma un ragionamento collettivo su quanto è in grado di sopportare il pianeta in termini di capacità di carico le future generazioni saranno costrette sicuramente a farlo. Ho ritenuto (perdonatemi, ma ci tengo molto; in questa Aula parlo spesso solo di infrastrutture, ma a volte ho voglia anche di andare oltre) di inquadrare il dibattito parlamentare odierno nel suo contesto globale, proprio perché dobbiamo aver presente che le cose di cui stiamo dibattendo, che richiedono azioni qui, nel nostro Paese, anche molto precise, molto settoriali e puntuali, in tale cornice internazionale, hanno questa complessità scientifica, hanno forti interrelazioni con le diverse azioni che accadono nelle diverse parti del mondo, hanno la necessità di tante azioni globali, perché non bastano naturalmente gli impegni, le carte e le parole, e soprattutto, hanno una straordinaria urgenza. Nel 1972 il MIT lanciò un allarme sui limiti dello sviluppo e indicò una preoccupante prospettiva di collasso se avessimo continuato a crescere nello stesso modo. Trent'anni dopo, nel 2002, rileva che la situazione si è notevolmente aggravata, ma che sicuramente ci sono anche dei segnali interessanti di attenzione e di azione, la consapevolezza

ritenere che quelli possano essere «la» soluzione del problema. Infatti, se riducessimo l'agricoltura tutta al servizio, per esempio, del trasporto e della mobilità,

e tenerli in equilibrio tra di loro. Una quota di carburanti deriverà sicuramente da produzioni vegetali, ma queste certamente non potranno sostituire interamente il complesso del petrolio,

il fatto di coinvolgere e rendere responsabili i cittadini che devono mutare i comportamenti, che devono essere d'accordo sulle scelte che li riguardano è una condizione essenziale di successo. Ancora, per la stessa sfida attore fondamentale è il mondo economico e industriale: e industriale: i Governi possono premere, i cittadini possono pretendere, le istituzioni mondiali possono scrivere, ma se il mondo industriale non accetta questa sfida credo che essa sarà persa in partenza. Certo, in Italia ci sono tendenze e contrasti all'interno del mondo industriale, in cui questa sfida, probabilmente proprio negli ultimi anni, è stata compresa nella sua complessità ma non pienamente accettata. Dentro Confindustria c'è chi parla di innovazione, di infrastrutture materiali, di biodiversità, di risparmio, di energie rinnovabili, di demolizione e ricostruzione, di risparmio del territorio, cioè con parole, linguaggi e idee innovative che guardano al futuro. però anche chi parla ancora di difendere il CIP6 (un sistema di incentivi sul quale tornerò), di carbone, di nucleare, di grandi opere autostradali e difende senza troppe sottigliezze

insieme quel confronto di merito e credibile per fare tutti dei passi in avanti, vedendo in questa materia un fattore di competizione, ma anche di equità e di giustizia sociale.

anche fare una riflessione sulle politiche dell'ambiente del centro-destra. Non voglio assolutamente negare - nel corso del dibattito di questa mattina ciò è emerso in diversi interventi - che all'interno del centro-destra vi siano persone, come l'ex ministro dell'ambiente Matteoli, che certamente hanno accumulato esperienze e idee e che si occupano di ambiente. Nella sua totalità, però, il centro-destra in Italia - diversamente da altri Paesi europei

La cosa che colpisce nel centro-destra italiano è che, diversamente da altri Paesi europei dove pure ha governato e governa il centro‑destra, la sfida ambientale non è stata assunta con quella forza e con quella capacità di iniziativa che è logico aspettarsi da forze politiche di massa come quelle presenti all'interno di quest'Aula. Dico questo perché in questo modo ci perdiamo tutti: non è soltanto un problema di destra o di sinistra. Vengo subito a dire che anche il centro‑sinistra ha delle arretratezze

passi in avanti, insieme alla nostra coalizione, ma chiediamo molto di più di quello che già è stato fatto - e nella nostra mozione lo abbiamo elencato - in materia di risorse, di fondi, di investimenti nel campo della sostenibilità. Ripeto: c'è certamente una netta, chiara inversione di tendenza, certi temi sono tornati nell'agenda politica quando negli anni precedenti erano sostanzialmente scomparsi, ma si deve e si può fare molto di più.

La cosa che colpisce ancora di più, però, è che, quando si parla di progetti come gli inceneritori (accade spesso anche per le grandi opere), uno degli argomenti fondanti che vengono invocati è che l'inceneritore rende, si paga da sé (a parte la cogenerazione), ma anche sul piano economico è un progetto che regge ampiamente sul mercato, quindi perché non farlo? Anzi, dobbiamo destinare almeno una quota in quella direzione. Quello che invece si scopre guardando all'ordine di grandezza degli incentivi (mi sembra

Bruxelles non dovremmo sostenere: quindi non stiamo contestando gli inceneritori (quello lo si fa mentre facciamo le politiche energetiche e le politiche dei rifiuti), ma stiamo contestando un sistema di incentivi

ad espanderla sta nel fatto che costa troppo, perché ovviamente ha una serie di costi di gestione assolutamente elevati. Quello che chiediamo è di riconvertire il sistema di incentivi da un sistema che

la richiesta che noi facciamo al Governo è questa (naturalmente c'è un disegno di legge all'attenzione della Commissione ambiente che poi sarà discusso noi chiediamo a tutti un grande impegno per superare questa situazione ed andare nella giusta direzione, anche ieri sono stati presi da parte dell'Unione degli impegni e noi saremo qui a fare in modo che questi impegni vengano rispettati.

e quindi una coerente politica d'attuazione del Protocollo di Kyoto, una coerente attuazione degli impegni che sono stati assunti anche in sede europea (Bruxelles

richiedono delle azioni e delle misure molto concreti per intervenire. Voglio porre tre questioni in particolare: un'attenzione fortissima alle città e ai pendolari, una forte innovazione del servizio, una revisione - com'è scritto nel programma dell'Unione - della legge obiettivo, almeno per tutta quella parte in cui prevede per il 60 per cento come infrastrutture nuove autostrade, che non farebbero altro che aumentare traffico e quindi CO2, emissioni e congestione. Signor

Bruxelles ci chiama - ed il Governo italiano ha avuto in questo un ruolo molto importante e positivo - a sfide ulteriori e rilevanti: quello che chiediamo al Governo è di essere all'altezza di queste sfide.

il Protocollo di Kyoto andrebbe letto nell'ottica di un più vasto contesto di azioni internazionali volte a fronteggiare i cambiamenti climatici del Paese, prendono le mosse dalla Convenzione ONU sui cambiamenti climatici adottata a Rio de Janeiro. Su questi cambiamenti climatici vorremmo avere anche, se è possibile, alcune certezze e conoscenze maggiori,

Gli impegni generali previsti dal Protocollo sono: il miglioramento dell'efficienza energetica; la correzione delle imperfezioni del mercato attraverso incentivi fiscali e sussidi; la promozione dell'agricoltura sostenibile; la riduzione delle emissioni nel settore trasporti; l'informazione rivolta a tutte le altre parti sulle azioni intraprese;

non trovano assolutamente alcuna applicabilità. I Paesi industrializzati si impegnano a ridurre le proprie emissioni entro il 2012, facendosi carico di maggiori responsabilità in considerazione dei bisogni di sviluppo economico dei Paesi in via di sviluppo.

Ora, sebbene la ratifica del Protocollo di Kyoto sia un atto dovuto, non si può tacere che lo stesso rappresenti un onere particolarmente gravoso per l'Italia rispetto ad altri Paesi europei.

e tale impegno risulta eccessivamente gravoso se si considera - è un fatto importante da sottolineare - che dal 1990 al 1998 le emissioni sono addirittura aumentate. Va altresì considerato che i Paesi firmatari non versano tutti nelle medesime condizioni. La Francia, per esempio, soddisfacendo il proprio fabbisogno energetico in gran parte attraverso la produzione di energia nucleare, non presenta livelli di emissione paragonabili a quelli del nostro Paese. Pertanto, deve sostenere e sostiene oneri oneri minori. Alla luce delle sopra esposte considerazioni, si può sostenere che la ratifica del Protocollo causerà verosimilmente notevoli problemi all'interno dei Paesi industrializzati, costretti a sostenere pesanti oneri,

anche se fonti autorevoli hanno stimato che tra il 1995 e il 2010 circa i tre quarti dell'incremento delle emissioni di anidride dalla Cina e dagli altri grandi Paesi in via di sviluppo già qui menzionati, come India, Indonesia e via dicendo. Pare, infine, opportuno opportuno richiamare gli studi e i convegni qualificati svoltisi in materia, sia in Italia che all'estero, i quali hanno sollevato non pochi dubbi circa la compatibilità

Nel corso di un recente convegno promosso da Confindustria, è emersa la preoccupazione per i costi di cui le aziende dovranno farsi carico per l'attuazione, appunto, del Protocollo, nonché le necessità di convogliare maggiori risorse alla ricerca e all'innovazione tecnologica, al fine di ricercare in tali contesti le soluzioni ai problemi connessi direttamente e indirettamente all'effetto serra. La recentissima approvazione del Piano nazionale di assegnazione delle quote di CO2 per il periodo 2005-2007 rappresenta, a mio parere, una vera e propria vittoria

causandone un forte rallentamento, se non addirittura il blocco. Per esempio, Energia Spa ha optato per il rinvio della realizzazione di un impianto sperando di poterlo fare con il prossimo piano 2008-2012. impianti che hanno un impatto negativo sulla concorrenza nel settore elettrico e sui prezzi dell'elettricità

non sono in grado di produrre energia elettrica a prezzi più bassi e con minore impatto ambientale, quindi il Piano non comporterà comunque alcuna riduzione

Inoltre, affinché l'Italia possa rispettare gli impegni prescritti dalla direttiva comunitaria 77/2001/CE, sulla promozione delle fonti rinnovabili, e e quelli connessi con il Protocollo di Kyoto, occorre incentivare soluzioni tecnologiche avanzate, ancorché commercialmente non competitive, riducendo gli incentivi non efficaci.

per la futura applicazione del Protocollo di Kyoto e per la relativa distribuzione delle quote di emissione sarà necessario far sì che la direttiva europea sull'*emission trading* trovi applicazione univoca in tutti i Paesi europei, recuperando le distorsioni che stanno emergendo nei mercati elettrici. Il diritto di emettere deve trovare corrispondenza nel diritto a produrre, in modo da stimolare l'efficienza produttiva e il miglioramento ecologico e ambientale e non precostituire immotivate posizioni di vantaggio tra le varie tecnologie.

Diversamente, il Protocollo di Kyoto rischia di determinare una sempre maggiore dipendenza dal gas naturale con evidenti rischi economici e di sicurezza del sistema. L'attuale portata del Protocollo di Kyoto non considera l'impatto dei Paesi «non Kyoto» che sono per la maggior parte i produttori di CO2. Questi ultimi attualmente già emettono più CO2 della somma di tutti gli altri Paesi. Appare pertanto illusorio affrontare gli obiettivi posti dal Protocollo limitandosi all'efficienza energetica di Europa e Giappone, che rappresentano una modesta frazione del problema. Occorre porsi il problema dell'Italia che si è autoimposta - come sempre siamo più realisti del re - obiettivi molto più onerosi rispetto ad altri Paesi dell'Unione, con la conseguenza di un'asimmetria nei confronti, per esempio, dei nostri amici tedeschi.

Signor Presidente, l'allarme clima, e ambiente è sicuramente una questione globale, non è un modo di dire. È la prima vera emergenza che riguarda tutti, senza confini senza confini che possano permetterci di dire: «Il problema non è nostro» o: «Il problema lo possiamo risolvere da soli». Proprio per questo motivo non si può affrontare demagogicamente il problema. Sono necessari grande realismo e grande senso pratico, cosa che talvolta rischiano di venir meno. Realismo vuol dire innanzitutto analizzare con serietà come intervenire, evitando di ritrovarsi a svuotare il mare con un cucchiaino. Realismo è l'opposto dei comportamenti che ci hanno portato ad uscire dal nucleare. Per questo è necessario intervenire su due filoni principali, distinti ma indiscutibilmente necessari. Innanzitutto con una politica di coinvolgimento seria, globale. I Governi devono operare per concertare, per responsabilizzarsi a vicenda, per capire che o si opera insieme o si rischia di lavorare per nulla. Questo non preclude, anzi impone un grande senso di autoresponsabilità; operare al proprio interno per essere virtuosi. Però essere virtuosi non significa essere autolesionisti: significa contribuire al miglioramento di un mondo che vorremmo consegnare alle prossime generazioni un poco meglio di come lo abbiamo ricevuto. E mi preoccupa sentire la senatrice Donati parlare di preoccupazioni per il carico umano del pianeta. Spero di aver capito male. La nostra è una visione diversa. L'uomo è una risorsa, non un problema! *(Applausi dal Gruppo* *UDC)*. L'uomo è al centro, deve tutelare l'ambiente per se stesso, non per l'ambiente! Nessuno ha intenzione di rinunciare al benessere acquisito; ma proprio questo il Governo deve agire al fine di incentivare i comportamenti virtuosi e, se si vuole essere polemici,

di educazione all'uso delle materie prime, all'uso dell'energia, con informazioni vere alla popolazione sull'efficienza di tutti i sistemi, attraverso la diffusione di stili di vita sostenibili e di conoscenze sui nuovi impianti.

in specifici Ministeri, compreso quello dell'ambiente, ma affidate direttamente ad una funzione di coordinamento generale che dovrebbe fare sintesi sotto la Presidenza del Consiglio. E non dimentichiamo l'impatto sul mondo della produzione perché, senatrice Donati, la via democratica all'ambiente non è quella della Cina. Un impatto che, vista la concorrenza sleale, si deve affrontare, ma non è sicuramente indolore proprio perché di globale non c'è solamente il clima, con i suoi problemi conseguenti, ma anche la competizione economica. Competizione senza regole (sempre a proposito di via democratica) che fa paura alle nostre imprese, specialmente a quelle medie e piccole. Tante aziende che economicamente fanno fatica a fare innovazione, tante aziende che culturalmente fanno fatica a guardante avanti, a guardare al cambiamento! Ma

numerosi casi hanno avuto la capacità di anticipare i tempi; molte hanno capito che l'ambiente può anche diventare economico, anzi un affare.

Probabilmente scandalizzerò qualcuno, ma non credo ai cambi repentini del clima per mano dell'uomo, così come non credo ai toni drammatici che da più parti vengono usati. Ci sono scienziati di fama mondiale, che hanno all'attivo innumerevoli scoperte, che la pensano in modo completamente diverso. diverso. Sono convinto, purtroppo, della nostra leggerezza di uomini: di uomini che si sono mossi con poca avvedutezza nella tutela dell'ambiente, di quello stesso ambiente nel quale l'uomo deve vivere.

Dunque, senza toni da catastrofe, impegniamo il Governo a continuare sulla strada di una seria politica di difesa dell'ambiente: continuiamo a lavorare per convincere tutti gli Stati del mondo ad impegnarsi con fatti concreti, concreti, per creare un clima politico globale. Dunque, diciamo sì all'attuazione del Protocollo di Kyoto e al rafforzamento della politica di ricerca, facendo del risparmio energetico una priorità, una sfida per tutti noi.

senza che questi vengano vanificati dai comportamenti poco virtuosi di coloro che, trovandosi in fase di crescita incontrollata e senza regole, continuano ad inquinare.

l'UDC intende praticarla ed è pronta a confrontarsi su questo nodo che, quando si esce dalle enunciazioni pure e semplici, è il vero nodo spinoso della politica.

fa sì che gli incentivi economici vadano, invece che alle fonti energetiche rinnovabili, a quelle assimilate (cioè a chi brucia rifiuti o utilizza i gas prodotti dalla lavorazione del petrolio).

È stato detto che lo stralcio dell'emendamento si è reso necessario per evitare l'ostruzionismo dell'opposizione, ma abbiamo visto stagliarsi le lunghe ombre del partito degli inceneritori. Un partito che non conosce partiti, ma solo il richiamo miope ed irresponsabile, socialmente pericoloso, del profitto immediato e degli affari facili, di quanti stanno cercando di accelerare i cantieri per accaparrarsi i fondi, di quanti minacciano, in una vergognosa opera di disinformazione, il rincaro delle tariffe della raccolta dei rifiuti (come a Torino, dove la società che vuole costruire l'inceneritore perderebbe 20 milioni di euro all'anno). Soldi dei cittadini, che dovrebbero finanziare le fonti di energia solare ed eolica e non, piuttosto, essere un sussidio dato alle aziende, in spregio alle normative dell'Unione Europea. Pertanto, dobbiamo fare, fare in fretta e fare la cosa giusta. In questi ultimi mesi - com'è stato sostenuto in moltissimi interventi è stato lanciato da più autorevoli parti l'allarme sul riscaldamento globale e sulla crisi ecologica del pianeta: se ne sono occupanti i *media* tanto intensamente da risvegliare la sensibilità, l'attenzione e la preoccupazione di un vasto pubblico. Il Quarto rapporto del gruppo intergovernativo sui cambiamenti climatici (IPCC) esprime come inequivocabile - cioè con una probabilità superiore al 90 per cento - il rapporto fra aumento della concentrazione dei gas serra, dovuto alla combustione delle fonti fossili di energia, ed il riscaldamento dell'atmosfera terrestre. L'impatto del riscaldamento globale riguarda l'alterazione delle piogge, la maggior intensità dei cicloni, le ondate di caldo, le piogge torrenziali, lo scioglimento delle calotte glaciali e dei ghiacciai alpini, l'innalzamento dei mari, il mutamento di complessi climatici regionali, la la diffusione di malattie prima confinate in fasce equatoriali e tropicali, la scomparsa di specie e ambienti naturali. Secondo l'IPCC, è necessario ridurre di almeno il 60 per cento le emissioni di gas serra entro il 2050, per evitare il crollo economico ed ecologico; secondo il WWF, il 2050 è la data soglia oltre la quale cominceremo a consumare il pianeta e non, piuttosto, i suoi prodotti. Se il livello di concentrazione dei gas serra continuerà ad aumentare al ritmo attuale, la temperatura media globale è destinata a salire, provocando lo scioglimento dei ghiacciai e l'innalzamento del livello del mare: non si tratta solo della fine delle nevi alpine, ma del rischio concreto, per almeno un miliardo di persone, di inondazione; ben due miliardi, invece, potrebbero essere inondati nel 2050, cioè un terzo della popolazione. A pagare saranno, com'è consuetudine del capitalismo, i Paesi e le popolazioni più poveri. Quello che ho letto finora, non è il catalogo di spettacolari effetti speciali di qualche film del filone catastrofista, ma sono previsioni di cui misuriamo già la portata descrittiva e realistica nel quotidiano. D'altronde, è di questi giorni l'allarme acqua e siccità lanciato anche nel nostro Paese. Abbiamo, perciò, ora, una grande ed essenziale responsabilità nei confronti dei e delle giovani e delle generazioni future: quella di consegnare loro questa terra, l'unica che abbiamo, in condizioni non irrimediabilmente compromesse. L'impegno deve essere mettere al centro delle decisioni e delle scelte le preoccupazioni per l'ambiente. Il nostro impegno deve essere, allora, quello di consegnare alle generazioni future una nuova razionalità economica, non fondata sulla inefficacia del mercato, sulla competitività e sul consumismo individualista, che generano iniquità sociale, sfruttamento del lavoro e della natura, non fondata, ancora, sulla crescita illimitata del prodotto. Serve, quindi, un cambio di paradigma di paradigma che possa mutare il sistema energetico nazionale e mondiale a partire da una strategia che nel medio periodo sia in grado di sviluppare l'impiego delle fonti rinnovabili di energia, la promozione del risparmio energetico, la trasformazione del sistema trasportistico. La riduzione di emissioni è obiettivo necessario, ma non può diventare l'alibi per riproporre ipotesi di rilancio del nucleare e impiego del cosiddetto carbone pulito, come invece è emerso dal G8 dello scorso luglio a San Pietroburgo: dentro questa logica, le energie rinnovabili svolgono soltanto un ruolo marginale piuttosto che rappresentare una priorità assoluta. Dobbiamo partire dalla riduzione delle emissioni di gas, lavorare per la sostituzioni delle fonti fossili di energia, ma avere mete ancora più ambiziose che hanno a che fare con la possibilità di costruire un mondo nuovo e migliore. Il 9 marzo l'Unione Europea si è impegnata ad una riduzione unilaterale delle emissioni di gas serra del 20 per cento rispetto ai livelli del 1990 entro il 2020 nonché ad un aumento della percentuale

entro il 2030 e del 50 per cento entro il 2050. In Italia, intanto, in assenza di una seria politica per rientrare negli obiettivi di Kyoto, le emissioni di gas a effetto serra hanno continuato ad aumentare. Nel 2003 le emissioni hanno superato i 577 milioni di tonnellate di anidride carbonica e nel 2004 si sono attestate attorno ai 583 milioni di tonnellate di anidride carbonica (fonte APAT). Se le energie rinnovabili sono il futuro, l'Italia è andata in direzione contraria, questo innanzitutto grazie all'eredità lasciataci dal precedente Governo che non è stato capace di cogliere la sfida economica e sociale che il cambiamento climatico comportava. Dal 1997 ad oggi il contributo delle energie rinnovabili è diminuito, passando dal 16 per cento del 1997 all'attuale 15,3 per cento. Nel 1990, anno di riferimento per il Protocollo di Kyoto, le emissioni erano pari a circa 520 milioni di tonnellate di anidride carbonica. Si è dunque registrato un incremento dell'11,1 per cento nel 2003 e del 12,2 per cento nel 2004. L'obiettivo di Kyoto è invece di tagliare del 6,5 per cento le emissioni registrate nel 1990 e dunque di ridurre le emissioni totali di gas a effetto serra a circa 486 milioni di tonnellate di anidride carbonica. Il *gap* da colmare entro il 2012 è dunque dell'ordine di circa 100 milioni di tonnellate di anidride carbonica. L'Italia non solo è il fanalino di coda dell'Europa, più lontano di tutti gli altri dall'obiettivo nazionale del 25 per cento di quota da rinnovabili sul totale del consumo energetico, ma è anche inadempiente rispetto agli impegni di riduzione delle emissioni di gas serra. Tra l'altro, le azioni in corso sono totalmente insufficienti a rispettare l'impegno assunto. Il nostro Paese è ancora un paese di sprechi di risorse, anche energetiche, eccessivamente dipendente dall'*import* energetico e dunque necessita di rispettare senza ritardo e dunque necessita di rispettare senza ritardo gli obiettivi europei posti per le rinnovabili, potenziando però al contempo l'efficienza energetica ed il risparmio. a raggiungere i più ambiziosi obiettivi europei delineati a Bruxelles, occorre eliminare qualunque sussidio ai combustibili fossili (anche se malamente travestiti da fonti rinnovabili, come

nello stesso periodo, la legge adottata nel 2.000 ha consentito attraverso le incentivazioni un aumento annuo di energia pulita di 3.000 megawatt, tanto che oggi si superano i 18.000 consideri che la cifra di 1.000 megawatt equivale alla metà della produzione di una centrale nucleare. La redditività degli investimenti è stata assicurata attraverso l'accesso una tariffa garantita per un periodo di 20 anni. I sovraccosti sono stati ripartiti su tutti i consumatori e sono di 5 euro a persona l'anno. Il settore ha creato 170.000 posti di lavoro mentre il cambiamento energetico ha consentito una diminuzione di emissioni di 7 milioni di tonnellate supplementari ogni anno, anno, risultati migliori che non quelli ottenuti con il mercato di scambio delle quote. Quindi, la Germania, la Francia, il sole della Spagna che è praticamente come quello dell'Italia, ci indicano che una strada è possibile, che si può fare, si deve fare, che è possibile farlo; ma bisogna agire subito, perché i prossimi anni saranno cruciali.

Signor Presidente, vorrei ringraziare innanzi tutto il presidente Matteoli per avere fornito al Senato l'occasione di questo dibattito con la presentazione della sua mozione, a cui sono seguite mozioni di altri colleghi. rivolgo è un ringraziamento non formale, così come credo che gli si debba un ringraziamento non formale per il lavoro che ha svolto durante i cinque anni di Governo nella scorsa legislatura. Questo dovrebbe bastare per ribattere alle contestazioni e ai rilievi che la collega Donati ha prima avanzato nei confronti della nostra parte politica.

vorrei focalizzare la mia attenzione su alcuni aspetti un po' differenti rispetto a quelli che ha trattato il dibattito. la mia piena adesione alle osservazioni del collega Possa, che mi pare siano state esposte in modo puntuale, documentato e con quell'atteggiamento che un uomo politico, ma anche un uomo di scienza, deve avere, cioè della capacità del dubbio e del ragionamento sui dati di fatto (quelli certi, quelli eventuali, quelli probabili e quelli ipotetici).

il primo è un diffuso catastrofismo che parte dalla stampa e dalla comunicazione, che su questi temi cerca la notizia, e la più eclatante possibile.

Ma questo riemergere del millenarismo apocalittico non nasce da sé e non nasce dalla scienza in quanto tale, ma dall'uso che delle acquisizioni scientifiche spesso la politica fa.

quale impedisce la riflessione ed il ragionamento sui fatti perché assume che esista una sola cultura pro ambiente e che questa sia composta da alcuni sillogismi che la scienza come tale non autorizza a formulare. Si parla, per esempio, del fatto che la comunità scientifica sarebbe convergente per il 90 per cento sulla tesi che l'emissione antropica di CO2 è quella rilevante a determinare gli incrementi di CO2 che si registrano.

poi sono diventato giornalista e quindi, come dire, l'intreccio tra le due cose mi trova particolarmente sensibile), intanto sa che non esiste la comunità scientifica: esistono scienziati, esistono laboratori, esiste soprattutto un fatto assoluto nella scienza, che è la contraddittorietà delle ipotesi rispetto ai fatti; e che nel contraddittorio e nella falsificabilità delle tesi (come ci ha insegnato Popper) si accertano le verità provvisorie che danno luogo a nuove ipotesi pronte ad essere falsificate, e quindi abbandonate, ovvero resistenti alla prova della falsificazione e quindi pronte a dare origine ad un nuovo quadro di conoscenza. scienziati e laboratori che operano in un ambiente di comunicazioni scientifiche (questo sì che esiste, perché la scienza ha come requisito il mettere a disposizione degli altri i propri risultati perché questi possano essere eventualmente falsificati) e c'è un dibattito aperto. Un dibattito che è aperto a tutt'oggi e, anche se gli scienziati che appartengono all'*International Panel* sono oggi in maggioranza propensi a credere alla tesi secondo la quale l'incremento della CO2 che registriamo è tutta, o prevalentemente, di effetto antropico, non vuol dire che tutta la scienza è giunta ad una conclusione certa e che condivide quella conclusione. Sarebbe saggio, da parte di chi ha responsabilità politica (la quale non comprende solo atti di Governo o decisioni, ma anche interlocuzione con i cittadini e capacità di informazione puntuale), che certi dati non venissero nascosti. Presidente, dalla lettura dei giornali sembra che il grosso della CO2 che il pianeta produce sia frutto dell'attività umana e che, invece, in natura la CO2 sia un elemento di scarso rilievo.

il mondo cerca di assumersi responsabilità condivise e globali rispetto a problemi che valicano i confini. Ma siamo sicuri che quanto disposto, con i relativi costi, porti a benefici misurabili? Qualche scienziato ha provato a valutare e ci sono degli straordinari grafici che indicano che, se non facessimo nulla, ci troveremmo in una situazione di crescita della temperatura globale stimabile con una certa curva, da qui al 2030, e che, se implementassimo tutto il Protocollo di Kyoto, otterremmo lo stesso risultato da qui al 2030. 2030. Qualcosa, evidentemente, non funziona. In che cosa non funziona? Intanto, nell'affermare che, se non si interviene subito, è il disastro domani. Grazie a Dio, il 2030 troverà altri a parlare di tali problemi in In secondo luogo, forse, le politiche che si vogliono adottare tendono ad essere irrilevanti rispetto al problema, ma enormemente onerose rispetto al sistema, il che non le fa vedere così vantaggiose, almeno a me.

come aveva scritto Umberto Eco negli anni Sessanta, come tra gli integrati che non vogliono nulla cambiare, contrapposto agli apocalittici che ci prospettano la fine del mondo prossimo. però che il Parlamento italiano, per la responsabilità che ha nei confronti dei cittadini e per quanto esso può influenzare la comunicazione, affrontasse questi temi in maniera molto meno assertiva evitando predizioni millenaristiche (scegliendo, cioè, un nuovo male assoluto che si chiama CO2). Signor Presidente, era ragazzo quando il Club di Roma, fondato da Aurelio Peccei,

Ora, chi leggesse quel rapporto, si accorgerebbe che la fine dello sviluppo era un titolo eclatante rispetto alla segnalazione di un problema che ci indicava come le risorse naturali debbano essere meglio utilizzate. Sono passati 30 anni, lo sviluppo non è finito ma si è moltiplicato a dismisura, e oggi il nuovo male sembra essere invece la CO2. Mi riservo di fare altre considerazioni in sede di dichiarazione di voto, ma vorrei indurre tutti i colleghi a riflettere. Questi problemi vanno affrontati con senso di responsabilità e il senso di responsabilità vuole che non ci sia un pensiero unico, che non si facciano accuse ingiustificate alle parti se sostengono tesi diverse e che non si dica al popolo una

il mio intervento desidera richiamare l'attenzione del Senato sottolineando l'importanza, una volta di più, del dibattito che stiamo facendo, sia pure in un momento abbastanza di riposo dei nostri lavori. L'argomento è molto importante non per pregiudizi di carattere dogmatico, ma per necessità di sviluppare un dialogo ed un confronto rispetto al quale i protocolli che sono stati adottati negli ultimi decenni ci spingono con forza e chiarezza e, se non fosse solo per i protocolli, a questo ci spinge ciò che accade sotto gli occhi di tutti noi. Il cambiamento climatico è nei fatti. Poi, certamente si discute di quali possono essere le sue ragioni ed è legittimo che ci siano opinioni contrastanti. Ci sono persino al riguardo della comparsa dell'uomo sulla terra: c'è chi afferma ancora che l'uomo sarebbe comparso 4.000 anni prima di Cristo e c'è chi afferma che sarebbe comparso, com'è molto probabile, per non dire certo, diversi milioni di anni prima. Quindi, figuriamoci se non è giusto e se non ci sono argomenti per discutere, come faceva poc'anzi il collega Stracquadanio, su quali siano le ragioni vere dei cambiamenti climatici in atto. Certo, però, che, se non bisogna essere allarmisti, c'è motivo di essere preoccupati e credo che da qui si debba partire. Ed è giusto che da qui partano i documenti che sono al nostro esame e che intendo sostenere, a cominciare dal documento presentato dai colleghi del Gruppo dell'Ulivo. Vorrei ricordare che negli Stati Uniti esiste un'organizzazione non governativa, il *Bulletin of the atomic scientists*, il bollettino degli scienziati atomici, che dal 1947 riporta il grado di rischio atomico del mondo su un quadrante simbolico, conosciuto come *Doomsday Clock*, l'orologio dell'Apocalisse. Le lancette calcolano i minuti che separano il mondo da una presunta, e naturalmente non auspicabile, mezzanotte atomica. Fissato inizialmente a sette minuti dalla fine, alle ore 15,30 ora italiana del 17 dicembre scorso, l'orologio è stato portato avanti di due minuti, dalle ore 23,53 alle ore 23,55. Mancherebbero cioè soltanto cinque minuti di tempo al pericolo di una catastrofe mondiale. Qual è la connessione con il dibattito che stiamo svolgendo oggi qui, visto che l'iniziativa del *Doomsday Clock* nasce come iniziativa antiatomica e quindi di pace?

dovuto soltanto a rinnovati pericoli provenienti da un riarmo atomico che si registra in alcuni Paesi del mondo, ma anche dalla considerazione dei pericoli rappresentati dai cambiamenti climatici. Gli scienziati indipendenti che si riuniscono nel bollettino di cui parlavo prima hanno valutato che gli effetti dei cambiamenti climatici possono essere considerati nel lungo periodo tanto pericolosi quanto quelli derivanti dall'uso, ripeto, non auspicabile, di armi atomiche. Può darsi che ciò non sia sufficiente a convincere tutti della necessità di intervenire in maniera anche drastica in questo campo, ma credo che ci sia più di un motivo per considerare attendibili le preoccupazioni in atto. Del resto, stiamo uscendo da un periodo invernale. Oggi siamo ancora in inverno, ma credo, che, al di là della temperatura di quest'Aula, che forse è l'unico posto in Italia dove l'inverno continua a manifestarsi, ormai non ci sia più nessuno nel nostro Paese che si comporta come se si fosse in inverno, a seconda naturalmente delle latitudini e delle circostanze. Qui a Roma siamo come in avanzata primavera. Le preoccupazioni che derivano da questo fatto non sono tanto nell'immediato (in primavera si sta bene, meglio che in inverno) ma rispetto a ciò che potrà avvenire la prossima estate. In qualità di componente della Commissione d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti, mi sono recato due settimane or sono in Campania, abbiamo incontrato il commissario straordinario Bertolaso, il quale ci ha detto di essere giustamente ed ovviamente molto preoccupato per la presenza di rifiuti nelle strade in questo momento, in vista dell'esplosione del caldo - ha detto e ha fissato, in questo caso, l'orologio della possibile esplosione del caldo, con preoccupazioni anche di carattere epidemiologico per la popolazione residente in quelle zone, risale, ripeto, a due settimane fa - quindi, di qui a pochi giorni, e non al mese di giugno, quando l'estate meteorologica dovrebbe iniziare. Sono segnali che certo possono essere considerati indizi e non prove, ma a fronte di questi ripetuti indizi ci sono valutazioni approfondite di scienziati e tutto questo deve essere tenuto nella dovuta considerazione. Certo, non possiamo forzare più di tanto l'economia globale e quella del nostro Paese, ma dobbiamo mettere in atto

possono essere definiti ecologici ma che possono anche essere considerati semplicemente di buonsenso e che forse appartengono molto più di quelli cui ci siamo abituati nei decenni trascorsi alle antiche tradizioni contadine, e non solo, delle nostre popolazioni. Non si tratta di tornare al buon tempo andato, ma di adattare a tempi diversi e situazioni diverse atteggiamenti di buon senso, considerando che la terra che ci è dato di abitare non rappresenta un bene indistruttibile in assoluto ma è qualcosa che deve essere conservato e difeso, naturalmente in funzione della generazione presente e anche - mi permetto di dirlo ‑ in modo particolare di quelle future.

che deve essere affrontato nelle scuole, nei luoghi di formazione, anche permanente, perché si acquisti una mentalità in grado non di valutare dogmaticamente, ideologicamente questioni che attengono la vita di tutti i giorni e di tutti noi, semmai, al contrario, di utilizzare criteri virtuosi e mettere in atto politiche adeguate. Spero che non sia il caso di ripercorrere testi letterali del passato, ma ricordo il manzoniano don Ferrante che, rifiutandosi di misurarsi con la realtà della peste, pensava

delle nostre conoscenze e soprattutto dei nostri comportamenti virtuosi in questo campo. *(Applausi

questa mattina in Aula sia stato importante e certamente ha messo a fuoco molte e varie tematiche. Il Governo non può che

politiche integrate miranti alla riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra. Non occorre in questa sede sottolineare le preoccupate riflessioni che in molte sedi scientifiche sono state avanzate e ricordare il fatto che finalmente questo tema stia entrando con più decisione nell'agenda dei Governi a livello mondiale.

La prima: un più incisivo impegno per lo sviluppo delle fonti rinnovabili; la seconda: un'efficace azione a sostegno del risparmio e dell'efficienza energetica; la terza: una limitazione degli incentivi per la produzione di energia alle sole forme non inquinanti; la quarta: l'introduzione di una programmazione energetica che miri a superare la dipendenza dai combustibili fossili; la quinta: il potenziamento degli strumenti di programmazione degli interventi per la riduzione dei gas ad effetto serra. Il Governo condivide queste sottolineature e, prima di esprimere il parere sulle mozioni presentate, presentate, mi compete solo ricordare ciò che il Governo ha fatto in questo periodo in cui ha avuto la responsabilità di governo del Paese, appunto per dimostrare che non servono solo le parole, ma servono soprattutto i fatti. Sul primo dei punti, quello riguardante un incisivo impegno per lo sviluppo delle fonti rinnovabili e sul secondo, che riguarda l'efficace azione a sostegno del risparmio e dell'efficienza energetica, vorrei ricordare che, con un insieme di strumenti principalmente contenuti nella legge finanziaria per il 2007, abbiamo messo a punto un pacchetto di interventi veramente imponente. Voglio ricordarne alcuni: la riqualificazione degli edifici, con un meccanismo molto forte di incentivazione per gli interventi che consentono di ridurre le dispersioni termiche, l'installazione dei pannelli solari e la sostituzione di vecchie caldaie con nuove ad alta efficienza; a favorire l'efficienza dell'industria, con detrazione fiscali atte ad incentivare l'acquisto e l'istallazione di motori a maggior efficienza; il pacchetto di interventi per la mobilità sostenibile, con la riduzione del carico fiscale per il GPL e l'incentivazione per la creazione di un parco-auto ecologico;

l'introduzione di un apposito fondo Kyoto con una dotazione di 600 milioni di euro per il triennio 2007-2009, che consentirà appunto di stanziare finanziamenti a tasso agevolato per i soggetti pubblici e privati che interverranno in questa direzione. Sono poi entrati in vigore i nuovi incentivi per il fotovoltaico, che certamente costituisce un sistema più efficiente di quello del passato per aumentare il contributo di questa fonte e anche per consentire un quadro certo, di sicuro stimolo per gli investimenti e l'innovazione tecnologica, creando le premesse per la costruzione di una filiera italiana dell'energia solare. Ricordo che il decreto elimina anche il tetto annuale che finora era stato previsto e fissa un obiettivo ambizioso per il 2016. È in via di potenziamento il meccanismo dei certificati bianchi; si potenzia e si rivede la modalità di incentivazione delle fonti rinnovabili: in questo caso lo strumento principale sarà

provvedimenti, in modo da poter predisporre un quadro organico di forme adatte di incentivazione delle fonti rinnovabili. intervenuti con l'incentivazione per la cogenerazione ad alto rendimento e abbiamo dato nuovo impulso alla bioedilizia attraverso il decreto legislativo n. Infine, voglio ricordare che viene avviato un progetto di innovazione industriale sull'efficienza energetica per la nascita e il radicamento di un'ecoindustria, con lo scopo di realizzare un'industria che utilizza meno energia nei processi produttivi e realizza nuovi prodotti capaci di rendere l'Italia più competitiva. Voglio qui ricordare che sarà Pasquale Pistorio il *project* *manager* che coordinerà lo *staff* per il lancio del primo progetto: riteniamo che questa scelta sia importante e che indichi anche la volontà di un'alleanza forte con il sistema produttivo del nostro Paese su questi temi. il terzo punto, cioè la limitazione degli incentivi per la produzione di energia alle sole forme non inquinanti, voglio riconfermare l'obiettivo del Governo, molto precisato, che si è espresso anche con la presentazione di un apposito disegno di legge destinato a migliorare la norma contenuta nella legge finanziaria del 2007, vale a dire il principio che gli incentivi alla produzione di energia

impianti, nel quadro delle sostenibilità del bilancio, debba avvenire attraverso un appesantimento della bolletta energetica di tutti i cittadini o debba trovare, più propriamente, un proprio finanziamento attraverso la tariffa che i cittadini che utilizzeranno

all'introduzione di una programmazione energetica che miri a superare la dipendenza da combustibili fossili, ricordo che i Ministri dello sviluppo economico e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare hanno deciso di costituire un apposito comitato interministeriale per la promozione della III Conferenza nazionale dell'energia e dell'ambiente; una conferenza finalizzata a definire una strategia nazionale energetica e ambientale, esaminando gli scenari a breve termine per superare l'attuale fase di emergenza del sistema energetico. altresì gli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili contenuti nel programma di Governo. Ricordo ulteriormente che il Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare ha a sua volta in previsione l'organizzazione di una specifica conferenza

ricordo che il Governo ha varato il Piano nazionale per l'assegnazione delle quote di emissione di gas effetto serra per il periodo 2008-2012, che attualmente è ancora all'esame della Commissione Europea. Il Piano prevede l'assegnazione di quote complessive coerente con gli impegni assunti. Il Governo sta lavorando alla preparazione della delibera CIPE di revisione delle linee guida per la riduzione dell'emissione di gas effetto serra, che costituirà il documento di programmazione per il periodo fino al 2012. Ricordo ancora lo stanziamento previsto nella legge finanziaria 2007 di un apposito fondo per il finanziamento delle misure finalizzate all'attuazione del Protocollo di Kyoto. Sulla base di queste riflessioni di carattere generale esprimo, quindi, il parere del Governo sulle mozioni presentate. Sulla mozione n. 65, a prima firma del senatore Ferrante, il parere è favorevole con la richiesta di una modifica riguardante il terzo capoverso, a pagina 5 del fascicolo. Si chiede di sostituire il testo con il seguente: «a valutare la possibilità di intervenire in modo da incentivare il risparmio dei consumi dei consumi elettrici «domestici», applicando tariffe ridotte in bolletta agli utenti che realizzano una diminuzione dei consumi pari almeno al 10 per cento all'anno precedente».

esistono impostazioni di politica economica ed anche energetica che tra di noi vedono una dialettica accesa in una differenza di valutazione. Tuttavia, penso che sia importante cercare di

di vista, le azioni che hanno svolto nel periodo in cui hanno avuto responsabilità di Governo. A mio parere, si dovrebbero lasciare da parte queste valutazioni perché ciò naturalmente richiederebbe da parte dell'opposizione di allora, che oggi è maggioranza, una serie di considerazioni sulle inadempienze che, a nostro avviso, si sono verificate, ma non è questo il punto che interessa. Chiedo allora di espungere dal ragionamento che viene fatto tutta una serie di considerazioni, che sono certamente sul tappeto della discussione politica e scientifica, sulla possibilità e sulla efficacia di azioni limitate alla sola iniziativa europea o allargata anche ad altri Paesi. chiedo, per poter esprimere un parere positivo, di voler accettare le seguenti modifiche. A pagina 7, al secondo capoverso, chiedo la sostituzione delle parole: «che non servono» con le seguenti: «che non sono sufficienti»; a circa metà pagina l'eliminazione della frase che inizia con le parole: «l'Europa può decidere di andare avanti»; al terz'ultimo capoverso l'eliminazione del primo periodo: «durante gli anni del Governo» fine a punto a metà della pagina 8 l'eliminazione del paragrafo: «secondo alcuni studi» fino al punto e virgola successivo; all'ultimo capoverso di pagina 8, dopo le parole: «potrebbero consentire una riduzione» aggiungere le seguenti: «considerevole delle emissioni di CO2con una attiva presenza di imprese italiane», eliminando tutto il periodo successivo; a pagina 9, al secondo paragrafo, dopo le parole: «rifinanziare il Fondo istituito presso la Banca Mondiale al fine di promuovere i progetti di cooperazione», cancellare

ha destinato al Fondo per lo sviluppo sostenibile 25 milioni di euro annui e che, all'interno di quello stesso Fondo, si prevede il finanziamento di progetti internazionali per la cooperazione ambientale sostenibile. Vorrei ricordare, inoltre, che il Ministero dell'economia sta attualmente predisponendo il provvedimento legislativo per autorizzare il contributo italiano, essendo l'Italia Paese donatore, al Fondo globale per l'ambiente, il Fondo multilaterale amministrato appunto dalla Banca mondiale. Infine, nel capoverso successivo il periodo si dovrebbe fermare al punto e virgola posto dopo le parole: «ma anche alla competitività delle imprese nazionali». Nell'ultimo capoverso, poi, si sottolinea l'opportunità di un intervento dello scorporo degli investimenti per l'attuazione del Protocollo di Kyoto dal Patto di stabilità. Naturalmente, il senatore Matteoli sa che la faticosa la riformulazione del Patto di stabilità si è conclusa senza la previsione di formule di scorporo di investimenti, quindi la possibilità di una attuazione dobbiamo riconoscere che può essere limitata. Tuttavia,

Sodano, il parere è favorevole con la richiesta di modificare il penultimo paragrafo di pagina 12, in questo modo: «prevedere gli opportuni interventi per aumentare l'efficienza e per ridurre le emissioni di gas a effetto serra degli impianti a carbone esistenti». Infine, sulla mozione 76, di cui è prima firmataria la senatrice De Petris, esprimo parere favorevole.

desidero prima di tutto ringraziare il Governo per l'attenzione riservata alla mozione presentata dal Gruppo di Alleanza Nazionale. Le modifiche che sono state richieste non stravolgono il senso della mozione da noi presentata, anche se la rendono meno efficace, perché è stato richiesto di cancellare alcune parti della mozione che mettevano chiaramente in risalto lo stato dell'arte.

C'è un aspetto, però, che reputo positivo. Su un argomento come questo, gradirei uscire da quest'Aula con le mozioni approvate, se non all'unanimità, a larghissima maggioranza,

L'aver citato le previsioni su una calda estate in un momento in cui la primavera è mite non ci autorizza a dire che è cambiato il clima perché notoriamente l'estate è calda e può essere più o meno calda e notoriamente la primavera è mite e può essere più o meno mite o più o meno lunga. Il punto, signor Presidente, è che certo modo di pensare, certo pensiero unico, è autoreferenziale e tutto tende a giustificare in base alla tesi che ha assunto. In qualche anno abbiamo avuto inverni miti e si è detto «è colpa del riscaldamento del pianeta», li avremo freddi in futuro e si dirà «è colpa dello scioglimento dei ghiacci che ci stanno portando masse di acqua fredda» o quant'altro. In sostanza, giustifichiamo a posteriori eventi nel breve tempo, parlando, invece, di fenomeni che hanno una prospettiva non storica, ma addirittura geologica. Se commettiamo questo errore culturale e in primo luogo scientifico, racconteremo

investimenti seri nel campo dell'innovazione, della ricerca e delle energie rinnovabili il sistema industriale italiano rimarrà tagliato fuori, non reggerà. Affermo con molta chiarezza che chi discute di competitività deve capire che oggi si deve avere il coraggio di accettare questa sfida fino in fondo oppure tutto l'apparato produttivo, che è già molto arretrato,

Siamo senz'altro favorevoli ad alcuni passaggi, che vedono i servizi pubblici essenziali - per esempio, l'acqua ancora di pertinenza delle piccole realtà comunali e degli enti locali; però, se vogliamo veramente affrontare questi argomenti

nonostante i continui sforzi per migliorare l'efficienza energetica, la domanda di energia ha registrato un incremento dell'8 per cento l'anno; le più recenti previsioni, invece, indicano un aumento del fabbisogno di circa l'1,5 per cento. Di conseguenza, in mancanza di provvedimenti adottati sulla base del riesame strategico di tutta la politica energetica, le emissioni di gas ad effetto serra

Alla luce di quanto sopra, dunque, mi chiedo questo: se vogliamo veramente ragionare di Kyoto, come possiamo parlare al contempo di sistema di parchi nazionali delle aree protette, della nuova normativa sperimentale sui farmaci, dell'azione di protezione per il benessere degli animali? Parliamo di argomenti seri e affrontiamo anche il problema, che viene ridiscusso, a livello europeo, da Paesi come la Slovacchia, il Regno Unito, la Bulgaria e la Romania, che hanno riaperto il dibattito della loro politica nucleare. Mi riferisco al fatto di riaprire il dibattito, tenendo presente che si è già svolto un *referendum*, in cui il popolo italiano si è dichiarato contrario. Chiedo solo di essere un po' realisti in quello che ci accingiamo a fare.

Siamo consapevoli della drammaticità dei problemi ambientali di fronte a noi; rifiutiamo un fondamentalismo ambientalista che non riconosce le componenti cicliche insite nei mutamenti climatici, alle quali, certamente, si aggiunge l'intervento umano come fattore potenziante, ma che non può essere considerato l'unico elemento del cambiamento climatico. Non dimenticate che nel secolo XVII si è verificata una miniglaciazione che ha mantenuto i propri effetti sino al secolo XIX e poi è venuta progressivamente meno; nel secolo XIV i sentieri attorno al Monte Rosa erano ampiamente trafficati, proprio perché era diverso il clima,

l'uomo è il soggetto cui è affidata la cura della terra e dell'ambiente. Un vero ambientalismo non può non vedere la centralità della persona umana, come, tra l'altro, è ricordato in un celebre contributo del professor Robert Spaemann: quello che chiamiamo natura è un certo equilibrio fra cultura e natura, non è la natura com'è uscita dalle mani di Dio; quella originaria non vi è più da nessuna parte, tranne, forse, in qualche angolo dell'Amazzonia. Apprezziamo, quindi, la posizione emersa anche dal recente Consiglio europeo: abbiamo bisogno di una politica europea che, con realismo, prenda, però, seriamente di petto i problemi ambientali, anche fuori da una visione che oppone la tutela dell'ambiente ai meccanismi di mercato. Dobbiamo lavorare per l'ambiente - ove possibile, insieme con il mercato - per farlo in condizioni di di maggior efficienza ed efficacia. Ci sembra di rilevare tale visione nelle prime due mozioni; crediamo che nelle seconde due vi sia ancora l'immagine di un ambientalismo in parte desueto, che non può servire da guida alla posizione del Governo italiano.

Signor Presidente, accolgo l'invito ad essere particolarmente sintetico per consentire all'Aula di esprimere un voto

favore dei CIP6 che, come ha spiegato l'ex ministro Matteoli, sostengono impropriamente ed improvvidamente fonti che rinnovabili non sono, contribuisce a sostenere i grandi gruppi industriali che in questo Paese hanno lucrato.

per mitigare e controllare gli effetti degli attuali mutamenti climatici. Tali mutamenti non possono, infatti, essere ignorati e vanno affrontati con senso di responsabilità e grande pragmatismo, tenendo peraltro conto di ogni opinione scientifica, anche se minoritaria, per evitare inutili allarmismi catastrofici che non sono utili, al pari di una ottusa indifferenza alla risoluzione del problema. Vanno parimenti affrontati su scala globale, per evitare che siano vanificati gli sforzi già fatti da italiani ed europei arrecando oltretutto inutili pregiudizi alla competitività del nostro sistema produttivo. È con questo spirito che Alleanza Nazionale voterà a favore delle mozioni a prima firma Matteoli e Ferrante, esprimendo viceversa voto contrario su quelle successive, palesemente viziate da una deriva ideologica che ne mina irreparabilmente l'equilibrio e la credibilità.

Il modo in cui l'Italia affronterà questo problema avrà perciò importanti conseguenze per il nostro futuro. Desidero dare merito al presidente Matteoli di aver suscitato il dibattito di oggi con la presentazione della mozione di cui è primo firmatario e a favore della quale preannuncio fin d'ora il voto favorevole di Forza Italia. Va innanzitutto chiarito che anche le più aggiornate conoscenze scientifiche, pur avvalendosi dei più avanzati strumenti di rilevazione e calcolo previsionale, offrono ben poche certezze sulle cause e sulla possibile evoluzione del riscaldamento climatico. Tra le certezze vi è il forte incremento nell'ultimo quarto di millennio della presenza di anidride carbonica nell'atmosfera e l'aumento della temperatura al suolo di circa tre quarti di grado nell'ultimo secolo. È anche certo che le attività umane immettono nell'atmosfera massicce quantità di anidride carbonica, ma grande incertezza vi è su quanto l'incremento dell'anidride carbonica sia dovuto al fattore umano, su quanto questo influenzi la temperatura e, soprattutto, su quanto potrà avvenire nel corso dei prossimi decenni e fino al 2100. Sappiamo, infatti, che i mutamenti climatici sono stati numerosi sul nostro pianeta: ogni studente o ex studente sa o dovrebbe sapere che solo negli ultimi 500.000 anni (una piccola frazione nella storia della vita sulla Terra) vi sono state quattro grandi glaciazioni. È meno noto che vi sono stati anche diversi periodi di decine di migliaia di anni in cui la temperatura è stata superiore a quella attuale, come del resto è accaduto per parecchi secoli intorno al 5000 e al 2000 avanti Cristo e ancora dopo l'anno 1000. le cause e difficilmente individuabili e isolabili: dai numerosi moti del nostro pianeta alle variazioni nell'attività solare e vulcanica o nella quantità di anidride carbonica nell'atmosfera, che è ancora oggi al 96 per cento di origine naturale. Il principale presupposto del Protocollo di Kyoto per la limitazione dell'immissione di anidride carbonica nell'atmosfera è perciò il principio di precauzione rispetto ai possibili danni di un prevedibile ulteriore aumento di queste immissioni. Accanto al principio di precauzione, vi sono altri elementi, assolutamente certi, che ci spingono ad una particolare attenzione alla politica energetica. L'Italia dipende in larga parte da fonti energetiche non rinnovabili, importate da aree politicamente problematiche o da Paesi che proprio negli ultimi anni hanno mostrato di usare la fornitura di energia come arma arma di pressione politica. Ogni riduzione percentuale dell'uso di queste fonti, che generano una grande quantità di CO2, è un beneficio certo per la nostra bilancia commerciale e la nostra sicurezza energetica. Noi sosteniamo, infatti, fortemente il risparmio energetico, a condizione che sia attuato nell'ottica dell'efficienza e non di un pauperismo utopistico ed inconcludente; sosteniamo la promozione e lo sviluppo di fonti rinnovabili, tenendo conto dei limiti di molte di esse; sosteniamo gli impianti di produzione di calore mediante energia solare e la cogenerazione. Auspichiamo, inoltre, una migliore informazione sulle possibilità offerte in questo campo dalla tecnologia e dagli incentivi pubblici. Il risparmio e l'efficienza energetica, che vanno promossi in generale, per la pubblica amministrazione diventano poi un dovere, poiché gli sprechi in questo campo riguardano il denaro richiesto al contribuente, con tributi anche molto pesanti, specie sotto questo Governo. Non è perciò tollerabile vedere edifici pubblici tenuti a temperature tropicali d'inverno o siberiane d'estate, oppure riscaldati anche durante i periodi di chiusura o mal coibentati, con le finestre spalancate durante la stagione fredda o per incuria o perché sovrariscaldati. La stessa cosa accade anche in estate quando anziché regolare meglio i condizionatori d'aria, vengono spalancate le finestre, anche perché molti non sanno che il condizionamento migliora anche la qualità, oltre alla temperatura, dell'aria. Su questo la pubblica amministrazione dovrebbe anche dare il buon esempio, a cominciare dalle scuole e dagli edifici delle principali istituzioni, inclusa questa. Sappiamo che su questo ci sono grandi margini di miglioramento. Vanno anche introdotte norme che incoraggino una maggiore efficienza nei condomini, incentivando o concedendo maggiore libertà ai singoli. Si sarà fatto un grande passo avanti nel settore pubblico, quando si mostrerà e applicherà la stessa cura che ogni famiglia responsabile pratica a casa propria, tra l'altro ampliando l'uso dei termostati, che in molti edifici

Un primo problema è quello dei costi. L'energia proveniente da fonti rinnovabili ha costi molto più alti rispetto a quella proveniente dal petrolio o dal metano. L'energia solare ed eolica funzionano, evidentemente, solo quando ci sono il sole ed il vento, cioè in periodi limitati e non prevedibili. A queste produzioni vanno perciò affiancati impianti di altro tipo pronti ad entrare in funzione quando non c'è sole o non c'è vento, ma che hanno costi anche quando sono fermi, e questo va tenuto nel debito conto. Secondo problema: i limiti quantitativi. Per quanti sforzi si facciano, le energie rinnovabili non potranno soddisfare che una parte minoritaria del nostro fabbisogno energetico. I risparmi potranno dare risultati importanti, ma non oltre certi limiti. Il richiamo a stili di vita più sobri ha un valore più che altro morale. Quella di un mondo felice che dimentica, o quasi, le automobili, le macchine e la velocità di spostamento, è un'utopia che si rispecchia in un passato dove la popolazione era dieci volte inferiore ad oggi, la stragrande maggioranza dell'umanità giaceva nella miseria, nell'incertezza, ed in condizioni di lavoro e di vita tali per cui si viveva in media un terzo rispetto ad oggi. I ricordi idilliaci di quelle epoche ci vengono da una minoranza di privilegiati che potevano permettersi di evitare e disprezzare il lavoro stremante dei toccava alla quasi totalità dell'umanità. Il terzo problema è chi dice no a tutto. L'adesione al Protocollo di Kyoto e le norme dell'Unione Europea impongono limiti all'uso di carburanti fossili e questo fatto è di per sé estremamente gravoso. A questo peso, per l'Italia si aggiunge il grave *handicap* di scelte avvenute in passato, quali la rinuncia all'energia nucleare, un'energia del tutto priva di emissioni di anidride carbonica, della quale si avvalgono la maggior parte dei Paesi europei, a cominciare da Francia e Germania, nostri vicini e amici, ma anche, soprattutto, concorrenti. Sappiamo poi quali furibonde opposizioni vengano suscitate quando si tratta di costruire centrali elettriche di qualsiasi tipo, incluse quelle idroelettriche - l'energia pulita e rinnovabile per eccellenza -, per non parlare dei termovalorizzatori, che, in parte significativa il 50 per cento), sono alimentati da biomasse rinnovabili, oltre a costituire un modo efficace di smaltire i rifiuti. Ma non basta: gli stessi soggetti dicono no ad opere come il collegamento ferroviario Torino-Lione, che potrebbe spostare su rotaia molto traffico stradale, che, come noto, è grande emettitore di anidride carbonica. Con questa politica si va certamente verso il declino, e con dubbi e scarsi risultati dal punto di vista delle emissioni di gas a effetto serra. Se davvero si vuole fare una politica efficace in questo settore, occorre dire basta ai fondamentalismi ideologici e, ad esempio, tornare a valutare l'opzione nucleare, la cui tecnologia e sicurezza ha fatto passi da gigante da quando fu abbandonata a seguito di un *referendum* che, in sé, non prevedeva affatto la sua cancellazione. quarto problema è il fatto che le limitazioni del Protocollo di Kyoto coinvolgono solo una parte dei Paesi di questo pianeta. Gli Stati Uniti, primo Paese per emissione di CO2, hanno ritenuto di non aderire, pur avendo messo in atto alcune misure che vanno nella stessa direzione. Diverso è il discorso della Cina, che secondo le più recenti stime starebbe per superare gli Stati Uniti in questa classifica: la Cina è stata esentata da ogni limite per quanto riguarda le emissioni di anidride carbonica e la stessa cosa vale per l'India, il Brasile e altri Paesi che, in genere, hanno assai poco riguardo per i rischi ambientali. Le istituzioni europee, che chiedono un grande sforzo ai cittadini e alle imprese per soddisfare gli impegni del Protocollo di Kyoto, hanno perciò il dovere verso i propri cittadini di usare ogni mezzo per far condividere il peso anche a Paesi che sono ormai grandi potenze economiche e nostri spietati concorrenti nella competizione globale. Di fronte a tutto questo, esprimo, a nome del Gruppo di Forza Italia, il voto a favore della mozione del presidente Matteoli, anche in continuità con la politica da lui messa in atto come Ministro dell'ambiente nel Governo Berlusconi. Sottolineo un ultimo fatto: di fronte a questo problema non si può avere un approccio catastrofista o impressionistico, ma occorre un approccio scientifico che non dia per verità assolute le opinioni di una parte della cosiddetta comunità scientifica, che in realtà non è una comunità, ma un luogo dove c'è ampio dibattito. In ultimo luogo, ricordiamo che il principio di precauzione ispira il Protocollo di Kyoto e va applicato anche nei confronti di misure così onerose da essere esse stesse un pericolo e, dunque, anch'esse vanno affrontate con precauzione e buon senso.

anche alla mozione presentata dall'ex ministro Matteoli, così come modificata secondo le richieste concordate con il rappresentante del Governo. Penso che trovare un'intesa ampia su temi come questo sia un fatto di per sé importante, tuttavia non sfugge, ascoltando questo dibattito, che permangono fattori di differenza non trascurabili. Vorrei che questo voto fosse per lo meno esplicitato in alcuni nodi che dovrebbero unire la gran parte di questa Assemblea. Fra questi grandi nodi c'è il cambiamento climatico, così come richiamato dal Protocollo di Kyoto, ricondotto a cause antropiche, cioè a causa delle emissioni di gas serra. Alcuni colleghi hanno richiamato - è noto nella storia climatologica del pianeta - che vi sono stati in epoche, sia lontane sia più vicine, altri periodi di cambiamento del clima.

solo su base regionale, sia pure ampia, ma starebbero coinvolgendo, o potrebbero coinvolgere, l'intero pianeta, con possibili e temuti esiti, per taluni probabili, di portata molto più ampia, anche in ragione della loro causa specifica specifica «prevalentemente antropica», che denota la sua anomalia. Nella storia del pianeta non c'è mai stato finora un cambiamento prodotto da emissioni generate dall'azione dell'uomo. Ciò non nega gli altri cambiamenti, ma dà una specifica e particolare connotazione a questo. Da qui, l'accordo sulla necessità di attuare misure incisive per fronteggiarlo; questo è il secondo punto che va sottolineato della convergenza, spero più ampia possibile, che si realizza in questo ramo del Parlamento. In merito alle misure, si osserva che un singolo Paese non può affrontare un cambiamento così globale: non bastano solo i Paesi industrializzati, bisogna coinvolgere anche i Paesi in via di sviluppo, a partire dalla Cina. Verissimo: il cambiamento con il quale ci misuriamo oggi è frutto dell'accumulo della concentrazione di anidride carbonica che si è anni. In questi 200 anni la responsabilità delle emissioni accumulate dai Paesi industrializzati è largamente prevalente. Ancora nel 2004, la somma delle emissioni dell'India e della Cina coincideva esattamente con le emissioni di anidride carbonica dei soli Stati Uniti. Si prevede che entro il 2015 le emissioni della Cina supereranno quelle degli Stati Uniti, ma anche a quella data la storia accumulata dalle concentrazioni di anidride carbonica sarà attribuibile, per la gran parte, ai Paesi industrializzati. Quindi, è giusto puntare, come dice anche la mozione Ferrante, al coinvolgimento dei Paesi di nuova industrializzazione e della Cina innanzi tutto, senza dimenticare la principale responsabilità che sta sulle spalle dei Paesi più industrializzati. In parole, l'impegno comune non deve servire a motivare il disimpegno di nessuno, tanto meno il nostro, tanto meno quello dei Paesi più industrializzati. Bene fa quindi l'Unione Europea a proporsi come traino dello schieramento per il cambiamento del clima e a puntare a fare delle politiche innovative in materia energetica, e non solo, un elemento di innovazione globale, oltre che di contrasto alla crisi climatica. Vorrei, in concreto, sottolineare tre punti delle mozioni. la necessità di riformare il sistema di incentivazione delle fonti rinnovabili, cui è connessa la revisione del cosiddetto CIP6. Infatti, nella misura in cui il vecchio CIP6 incentivava con risorse pubbliche sulla bolletta pubbliche sulla bolletta fonti non rinnovabili, è evidente che avevamo meno risorse per incentivare le fonti rinnovabili stesse, che devono essere invece un pilastro della politica del Protocollo di Kyoto. sollecitare un programma nazionale che porti ad un rapporto sul cambiamento climatico in Italia. Sappiamo poco di ciò che sta già accadendo. Ci rendiamo conto che c'è una crisi idrica in molte aree, che ci sono pericoli di aridificazione, ma, in vista della Conferenza sull'energia, ci serve un rapporto Stern italiano per capire cosa sta accadendo, cosa può succedere; non solo quanto costano quanto costano le misure (e non ci saranno pasti gratis), ma quanto ci costeranno le mancate misure anche in Italia. Infine, sulla Conferenza energia-clima, apprezzo che il Governo ci comunichi che ci sarà una Conferenza